Signor Presidente, signor Vice Ministro, signor Sottosegretario, nel prendere la parola in questo strano e delicato dibattito, intendo esprimere la mia personale gioia per il ritorno alla libertà e alla famiglia del bravo e coraggioso giornalista Daniele Mastrogiacomo, selvaggiamente percosso,

Alla stessa pena era stato condannato, infatti, l'afghano che si era convertito al cristianesimo nella confessione luterana. Capisco che per i cattolici democratici dell'Ulivo il fatto che questi si fosse convertito alla confessione luterana non lo destinava a essere tutelato; ma per me, che sono *teocon* ma ecumenico, il principio è lo stesso. E intendo qui, anche a motivazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno che ho presentati, ringraziare chi ha il merito di questo esito non infausto della pericolosa vicenda. Anzitutto ringrazio i signori talebani, che anche per questo, oltre che per essere in Afghanistan il principale soggetto politico, insieme a quello che viene ingiustamente chiamato movimento terrorista, il forte e vittorioso movimento di Rivincita islamica Al Qaeda, in contrasto con le forze della NATO, si sono largamente meritati di sedere al tavolo della prossima conferenza internazionale di pace che sarà indetta dal Consiglio di Sicurezza, come ha proposto il segretario nazionale dei Democratici di Sinistra con il mio pieno plauso. Infatti, quando si fa una conferenza di pace al tavolo siedono gli avversari e non i Paesi vicini. Il secondo ringraziamento va al medico, dottor Gino Strada che è meritoriamente riuscito nelle sue iniziative che hanno avuto successo, in forza della fiducia che in questi anni egli si è acquistato (anche con i soldi del Ministero degli affari esteri), presso i signori talebani e il forte e finora vittorioso grande movimento di Rivincita islamica Al Qaeda, con la sua ferma e sprezzante opposizione e gli insulti rivolti alle unità militari italiane contro le iniziative dell'ONU e della NATO che hanno portato all'invasione dell'Afghanistan (contro la quale io ho sempre votato, così come sempre ho votato contro le operazioni in Iraq), al rovesciamento del Governo talebano di Kabul (responsabile, tra l'altro, di aver sconfitto l'Armata Rossa

alla guerra attualmente in atto, fortunatamente non più con la partecipazione italiana, perché l'Italia si è sganciata infine di fatto dai vincoli dell'Alleanza atlantica. Il ringraziamento va poi all'intelligente politica del ministro degli affari esteri Massimo D'Alema per avere ottenuto il via libera, dato dalle amministrazioni americana e britannica al Governo fantoccio di Karzai, alla liberazione di cinque alti dirigenti del movimento dei signori talebani; per avere compreso che solo un amico dei signori talebani e del potente movimento di Rivincita islamica Al Qaeda, poteva ottenere la liberazione dell'arrestato;

Lo si deve ringraziare per avere avuto il coraggio di prendere la delicatissima decisione di riconoscere politicamente i signori talebani e, indirettamente, il potente movimento, ingiustamente chiamato terrorista, di Rivincita islamica Al Qaeda, e anche per avere «stoppato» con decisione, con la sua clamorosa visita a piazzale Clodio, con decisione le improvvide iniziative della magistratura romana che avrebbero potuto portare anche all'esecuzione

sarebbe ingiusto. Mi auguro che il Ministro torni a piazzale Clodio. Ci fosse stato Massimo D'Alema al posto di Enrico Berlinguer al momento del rapimento di Aldo Moro! In fondo che cosa chiedevano le Brigate Rosse, se non il riconoscimento politico che oggi il Governo ha dato ai signori talebani e al suo alleato, il potente movimento di Rivincita islamica Al Qaeda? Ma che cosa chiedevano le Brigate Rosse se non la scarcerazione di due o tre combattenti della Resistenza incompiuta - come loro la chiamavano - e per di più malati, che nulla erano rispetto ai cinque grandi *leader* politico-religiosi-militari del grande movimento di resistenza armata, culturale e religiosa dei signori talebani e di Al Qaeda? Ma dov'eri allora, Massimo D'Alema? Ah, se ci fossi stato tu, allora! Certo, ma quelli erano i tempi modesti, vili e corrotti di Giovanni Leone, di Giulio Andreotti, di Arnaldo Forlani e di Francesco Cossiga, i cosiddetti «uomini della fermezza», di cui poi due accusati di corruzione,

Ah, se ci fossi stato tu, Massimo D'Alema! Io non mi sarei svegliato per due anni urlando: «Ho ammazzato Aldo Moro!», a me, Giulio Andreotti e Zaccagnini sarebbe stata risparmiata l'accusa infamante di «assassini», rivoltaci dalla famiglia - lo comprendo e la perdono - di Aldo Moro. Erano i tempi tristi di uno Stato debole e di un Governo debole. Erano i tempi tristi di un partito debole e trasognato come il Partito comunista italiano, unito in questa immorale e antiumana linea della fermezza. Non erano i tempi gloriosi di oggi, quelli attuali, di un Governo degli onesti, forte e deciso, pronto a muoversi, giustamente, per la salvezza di un uomo, senza dover ricorrere, come a quell'epoca, a sedute spiritiche.

vogliamo ritirarci dall'Afghanistan. Ma vogliamo paragonare il pericolo costituito da Silvio Berlusconi, che ha capito che prima se ne va, meglio è, al pericolo di Al Qaeda? Ma è molto maggiore il pericolo di Berlusconi! Ma per carità! E chi se ne fotte del popolo di Vicenza! Dall'altra parte c'è il pericolo di Berlusconi. Le trattative con i signori talebani, il nemico non certo nostro, questo sia chiaro, ma della ridicola ed in sé divisa e divergente organizzazione della NATO? Solo il presidente Andreotti ed io abbiamo

se le truppe canadesi che si trovavano in un pasticcio in Afghanistan hanno chiesto l'aiuto delle truppe tedesche e queste glielo hanno rifiutato. Quando in Kosovo - io c'ero - le

teorico cinese della guerra e dei conflitti Sun Tzu: «Se il nemico non lo puoi battere - e noi non possiamo battere i talebani per il motivo molto semplice che non li combattiamo - accordati con esso». Ma un forte ringraziamento deve andare anche al ministro della difesa Arturo Parisi, ed è doloroso che nessuno ci abbia pensato. Egli, dopo la costituzione del Governo di centro-sinistra, è riuscito, con la piena e leale collaborazione delle alte autorità militari, a mutare il carattere di operazione militare della presenza di unità delle Forze armate italiane in operazione di pace a carattere umanitario, anche a indirizzo agricolo e, a ben vedere, silvano (signor Sottosegretario, le sarei grato se lei volesse dirmi se sono 11.000 o 15.000 - secondo un comunicato del vostro Ministero - le piantine messe in opera; e mi meraviglio che non abbiate detto quante sono le scatole di gallette di tonno e di carne che avete distribuito), facendo ad esse, assumere progressivamente una posizione di crescente neutralità ed equidistanza tra i signori talebani, i signori tribali della guerra e il forte e vittorioso movimento, ingiustamente chiamato terrorista, di Rivincita islamica Al Qaeda, da un lato, e le forze combattenti della NATO, dall'altro, dalle quali ultimamente le nostre Forze armate si sono definitivamente sganciate e profondamente differenziate. Proprio per confermare e canonizzare in precise norme di legge l'indicato mutamento del carattere della presenza delle unità delle Forze armate italiane in senso non più militari, ma di pace a carattere umanitario, anche ad indirizzo agricolo e - secondo il comunicato del Ministero della difesa - a indirizzo prevalentemente silvano Certo eviterei di andare a costruire chiese cattoliche che poi dobbiamo demolire. In proposito bene ha fatto il Ministro a richiamare - secondo il comunicato del Ministero della difesa - l'incauto portavoce che l'aveva dichiarato e che credo verrà duramente punito.

dal controllo operativo della NATO, comandi centrali

e sono sottratte anche - salvo che non vengano cambiati - agli indirizzi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Perché non possiamo disobbedire alle Nazioni Unite? E se le Nazioni Unite vanno contro l'articolo 11

ha fatto il possibile: ha raddoppiato la base di Vicenza, dove si è rischierata, com'è noto, la 173a Brigata, che serve per andare a fare operazioni fuori area; ha rafforzato la base di Aviano, da dove sono partiti, insieme ai nostri,

ho assistito al consenso dato dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro degli affari esteri perché si scatenasse il bombardamento della Serbia e di Belgrado! C'ero, l'ho sentito con le mie orecchie: «Se proprio è necessario, andiamo.» Non dimentico quando Massimo D'Alema, con il giubbotto dell'Aeronautica militare, a Gioia del Colle passò in rassegna gli equipaggi dell'Aeronautica militare e della Marina militare, la prima volta che la Marina militare intervenne, per ringraziarli per il contributo dato a piegare Milosevic con trentacinque giorni di bombardamento, che hanno colpito obiettivi militari e civili. Questo i militari non lo dimenticano e per questo hanno grande rispetto, come ce l'ha l'America, per Massimo D'Alema.

Voterò, invece - e mi dispiace per gli amici della Lega - contro gli emendamenti e gli ordini del giorno che mirano a dotare di un più potente armamento le unità militari italiane, perché il Capo di stato maggiore della difesa, come ieri riferito a «Porta a Porta» dal vice Ministro, ha dichiarato che il leggero armamento di cui essi sono dotati, che è esattamente uguale a quello dei reparti mobili della Polizia di Stato e dei battaglioni mobili dell'Arma dei carabinieri, è assolutamente soddisfacente e forse anche eccessivo. a che servono gli autoblindo, signor Sottosegretario; per piantare gli alberelli? E a cosa servono gli autoblindo se dobbiamo distribuire scatole di gallette, di tonno e di carne? Non servono a nulla. Teniamo poi presente che i militari si possono far male. Andiamoci piano con gli armamenti. Si provvederà a dotarli di più pesanti armamenti quando, in nome della pace, dovranno impegnarsi a difendere i signori talebani, i signori tribali della guerra e il forte e vittorioso movimento di Rivincita islamica Al Qaeda dall'aggressione delle forze NATO. Signor

e fare un bilancio sulle pratiche di partecipazione di contingenti militari in missioni internazionali di pace. Questa strategia è andata affermandosi di pari passo con il principio della «responsabilità di protezione», ovverosia dell'impegno degli Stati sovrani a intervenire in aree colpite da conflitti o anche preventivamente in caso di gravi violazioni di diritti umani. La *responsibility* *to* *protect* oggi è uno dei cardini fondamentali del sistema delle Nazioni Unite e, quindi, autorizza anche una maggiore riflessione rispetto al buon esito di missioni a cui l'Italia ha partecipato finora; non soltanto l'Afghanistan, ma anche il Kosovo, le missioni nei Balcani, le missioni nel Corno d'Africa e altre oggetto di questo decreto. Quindi, la prima considerazione che vorrei svolgere è la seguente: sarebbe opportuno e utile effettuare una disanima concreta della pratica dell'ingerenza e dell'interventismo umanitario per comprendere se, spesso e volentieri, lo strumento militare non abbia preso il sopravvento rispetto a quello della politica e se queste missioni che dovrebbero essere di pace e, quindi, avere un combinato disposto di vari strumenti, alla fine non siano missioni militari con obiettivi di stabilizzazione di pace. pace. È un elemento che - a mio parere - forse è stato fin troppo poco sottolineato nella discussione che abbiamo avuto negli ultimi anni, in particolare sull'Afghanistan e non solo. Per quanto riguarda la questione dell'interventismo umanitario e, quindi, dell'uso dello strumento militare per promuovere la democrazia e i diritti umani, una delle questioni che oggi passerà sotto banco, sia

ci sono migliaia e migliaia di civili, vittime di scontri militari, e c'è la difficoltà del Consiglio di Sicurezza di intervenire con gli strumenti del diritto internazionale, da cui deriva il rischio di interventi unilaterali che sono assolutamente inaccettabili, sia nelle modalità che negli scopi finali. Eppure, il Darfur oggi non è al centro della nostra attenzione, dimostrazione che il principio dell'ingerenza dell'intervento umanitario spesso viene usato in maniera selettiva e va a pregiudicare anche uno dei perni fondamentali delle legalità internazionali: i diritti umani sono universali, indivisibili

La differenza che esiste tra la missione in Libano e quella afghana è fondamentalmente questa: troppo spesso sentiamo parlare della missione ISAF come di una missione ONU. Non è una missione ONU, ma una missione NATO, che a avuto una legittimazione *a* *posteriori* da parte della Nazioni Unite;

La NATO, invece, in Afghanistan ha deciso di scaricare su quel popolo la responsabilità di garantire la sopravvivenza stessa dell'Alleanza. Questo non lo possiamo accettare, perché pensiamo che oggi il dibattito sull'Afghanistan debba essere improntato sui bisogni veri di quel popolo, e non sulla necessità di consolidare un'alleanza che forse ha fatto il suo tempo o, certamente, di restituire quel popolo nella morsa dei talebani. talebani. Lo sforzo che oggi vogliamo compiere come pacifisti radicali e convinti, ma anche pragmatici nel nostro pacifismo, è proprio quello di fare un salto di qualità nella discussione. Non vogliamo più accettare la polarizzazione tra chi ci dice che la NATO debba essere il fine ultimo della nostra presenza in Afghanistan e chi invece sostiene che mettere in discussione quello strumento militare possa equivalere a restituire il popolo afghano alla dittatura dei talebani. Noi vogliamo una terza via: stiamo ridiscutendo anche di alcuni fondamenti dell'approccio pacifista alla politica internazionale. Pensiamo che oggi l'iniziativa assunta dal Governo possa rappresentare una via d'uscita diplomatica e negoziale. Dobbiamo capire, negoziale. Dobbiamo capire, quando parliamo di talebani, che non si tratta di un insieme omogeneo: ci sono talebani ispirati dal Pakistan, talebani che rappresentano la genuina opposizione e anche lo sconforto delle popolazioni locali afghane. Vi sono anche delinquenti e signori della guerra che magari fanno parte del Governo Karzai. allora necessario costruire una strategia che porti ad una conferenza internazionale. Guardate che con i talebani o ci si tratta o si pensa di annientarli tutti; quest'ultima ipotesi significherebbe inimicarsi tutto il popolo afghano. Allora la soluzione non ci sarà e i nostri saranno visti come un obiettivo primario di tipo militare. vediamo la conferenza internazionale come un processo e non come un evento; chiediamo al Governo di essere conseguente, di rafforzare la cooperazione civile, di andare incontro ai bisogni primari della popolazione afghana, di assicurare giustizia e verità per i crimini compiuti dai talebani e anche dopo e, soprattutto,

è stata una giornata abbastanza densa di impegni e di interessi. Questa mattina abbiamo sentito,

che verrebbe voglia di aprire adesso una discussione sulle dichiarazioni che ha fatto il presidente Cossiga, che sicuramente meriterebbero più attenzione

Presidente, ci viene posto un testo nel quale si dice cosa deve fare il nostro Paese d'ora in poi nei confronti dell'impegno militare sugli scenari più o meno di guerra.

Il guaio è che noi dovremmo dare una risposta unica ad un quesito che, di fatto, sottende due domande. La prima domanda è se noi dovremmo continuare a rimanere in Afghanistan, cioè se dovremmo continuare a garantire la pace in quel Paese, ad evitare recrudescenze, ad evitare che il Paese ripiombi nel buio dal quale è stato levato; levato; se dobbiamo rimanere con la comunità internazionale per bloccare un terrorismo senza volto, che, quando arriverà nei nostri Paesi, non riusciremo più a combattere, mentre sappiamo che lì si sta organizzando, addestrando, ingigantendo. A questa prima domanda non v'è dubbio che bisognerebbe, per senso di Paese, per spirito non dico di Nazione, ma di corresponsabilità che dovrebbe toccare ognuno, rispondere di di sì. Abbiamo però una seconda responsabilità. Chi c'è in quel posto? Abbiamo mandato circa 2.000 militari, 2.000 soldati italiani.

le sue parole - e per distribuir gallette probabilmente l'attrezzatura di cui dispongono è più che sufficiente. Ma noi sappiamo una cosa: tutti i Paesi hanno servizi di *intelligence*, tutti i Paesi presenti sullo scenario di guerra hanno informative che ci sarà un inasprimento della lotta e ci sarà una controffensiva da parte talebana. Lo sappiamo anche noi; e sappiamo che abbiamo dei militari inviati - mi si passi la metafora - d'estate con dei calzoncini corti, mentre adesso siamo alle porte dell'inverno.

la situazione nella quale si trova il vigile, che deve soltanto regolare il traffico, per cui basta forse uno sfollagente o un fischietto. Lì, secondo noi, i nostri militari devono avere tutto ciò che è necessario per affrontare tale momento. I nostri militari hanno tutto ciò? Hanno una strutturazione, mezzi idonei e attrezzature adeguate? No,

e lo dicono i generali dell'Esercito uditi ieri in Commissione difesa, che affermano addirittura che i mezzi di cui dispongono i nostri militari hanno un grado di efficienza che loro valutano del 60 Non conosciamo i parametri di giudizio ma suppongo che il 60 per cento sia un livello poco più che sufficiente. Con un parco mezzi così inefficace e insufficiente,

in Aghanistan, solo questo ci deve far dire che dovranno rimanerci anche domani», con tutte le situazioni che conosciamo e che stanno mutando in peggio e a rischio per i nostri militari?

Non credo che sia una richiesta così rivoluzionaria o stravolgente, ma se il Governo non accetterà che i nostri militari siano in quel posto con le dotazioni necessarie al momento noi non potremo irresponsabilmente dire che voteremo a favore di questo provvedimento.

contesti nei quali il migliore degli eserciti non può vincere: la Francia in Indocina, gli Stati Uniti nel Vietnam, l'Unione Sovietica in Afghanistan, oggi l'Iraq ed ancora l'Afghanistan. Pantani nei quali gli eserciti regolari affondano. Oggi nessun analista serio sosterrebbe che la presenza militare internazionale in Afghanistan sia vincente: poche truppe, nel nostro caso forse, come è stato già accennato, anche male armate. Noi mettiamo inutilmente a rischio la vita dei nostri soldati. In ogni caso, non si ottengono risultati mandando eserciti in in un Paese dominato dai signori della guerra e dell'oppio, con un apparato statuale praticamente inesistente, che non durerebbe più di pochi giorni senza la gruccia della presenza militare. Aggiungo che non si mandano truppe a sostenere un regime che nella sua Costituzione riconosce centralità alla *Sharia*. Per un caso della mia vita ho vissuto negli Stati Uniti gli anni più duri della guerra del Vietnam: ero un giovane studente alla facoltà di legge dell'università di Harvard. Ho visto amici fuggire all'estero per sottrarsi alla leva;

Da loro ho imparato, partecipando alle loro veglie, alle loro manifestazioni e alle loro proteste, che le guerre sbagliate non si fanno mai, in nessun caso. Da questo punto di vista, il mio voto sull'Afghanistan non potrebbe essere che negativo. Ma c'è un'altra-assorbente-considerazione. Qualche giorno fa, in Gran Bretagna, 80 componenti della Camera dei Comuni Comuni appartenenti alla maggioranza hanno votato contro il Governo sul riarmo nucleare, sulle prospettive, appunto, della pace e della guerra. Senza il concorso necessario dei conservatori, il Governo Blair non avrebbe ottenuto il positivo vaglio del Parlamento. Ebbene, noto che nessuno ha protestato, ha alzato lamentele, ha prospettato dubbi o ha chiesto che il Governo si dimettesse. Nel tempio del bipolarismo nessuno si è turbato per un voto in cui la maggioranza si è avvalsa del concorso necessario dell'opposizione. Potremmo fare lo stesso. E invece no. È stata inventata una teoria costituzionale per cui il voto *bipartisan* presuppone l'autosufficienza della maggioranza.

tesi evidentemente funzionali non già ad un corretto e razionale funzionamento delle istituzioni, ma alle tensioni e ai rapporti di forza interni alla coalizione di maggioranza e a quella di opposizione; tesi che vengono da un bipolarismo malato e, come mi capita spesso di dire, paranoico. Ciò che non si coglie è lo stravolgimento del tessuto costituzionale che ne deriva, tessuto che è e rimane quello di una forma di Governo parlamentare. come non si coglie la riduzione forzosa della capacità di rappresentanza del Parlamento, che non esprime affatto il sentire ampio e forse prevalente del Paese contro la guerra Il paradosso per me è che il mio voto negativo potrebbe essere quello che - decisivamente - pone i numeri della maggioranza sotto quella soglia, pur di fantasia. E potrebbe in tal modo contribuire all'attacco ulteriore alla Costituzione. Per questo voterò sì. Il mio voto favorevole, signor Presidente, non è a questo Governo o alla sua scelta politica, che non lo meritano. Assolutamente dissento: non si esporta la civiltà occidentale, tantomeno con le armi. E se fosse esportabile chiederei che venisse esportata in qualche sobborgo metropolitano molto più vicino a noi, in una delle nostre città. Questa è una guerra inutile e sbagliata dalla quale bisogna uscire. Il mio è un voto per la Costituzione della Repubblica, cui va la mia fedeltà molto prima che a questo Governo e a questa maggioranza. Il mio voto favorevole manifesta il rifiuto ad essere strumento, contro ogni mia diversa intenzione, di una lettura stravolgente della nostra Carta fondamentale, che la indebolisca ancora, aggiungendo danno ai molti già fatti. Un voto per la Costituzione repubblicana: questo è il solo ed esclusivo significato del mio assenso.

e forse ho anche un po' più di carità di patria. Ecco perché non affonderò il coltello nelle contraddizioni che sono dentro questa situazione politica, che non è quella iniziale ed è quella nella quale in questo momento viviamo. il mio amico senatore Zanone, a ricordarne la genesi: del resto nei documenti che ci vengono consegnati dagli uffici del Senato è scritto come è nata questa iniziativa, perché è nata, nata, chi ha creato il terrorismo esportato in America, quando tutti eravamo americani l'11 settembre, quello che appena il giorno dopo

personale e internazionale attraverso gli strumenti difensivi della NATO - e le decisioni che successivamente sono state assunte contro il terrorismo. È cambiato qualcosa da allora, onorevole rappresentante del Governo? Il terrorismo che ha nutrito Al Qaeda in Afghanistan, quello contro il quale ci siamo mossi insieme al consorzio internazionale, con il patrocinio, il sostegno e la deliberazione conforme delle Nazioni Unite, è cambiato o no? Questo è il problema che dobbiamo affrontare, per chi si pone in buona fede di fronte all'esigenza di allora e alla permanenza di oggi. Non si tratta di continuità o discontinuità, si tratta di quella che un tempo veniva chiamata coerenza. Non so se ora il termine possa essere più usato, qui o altrove. Parlo della coerenza rispetto agli impegni assunti,

È un esercito nascosto, che appare e scompare, e da questo punto di vista è anche più pericoloso. La differenza, fra le guerre di un tempo e quelle di oggi, per fortuna,

che ci sia l'aggressione alle spalle, che avvenga qualcosa mentre si circola per strada, che si determini un comando a distanza, da parte di chi è vile, o un comando più da vicino, da parte di chi è coraggioso, testimone della sua fede.

pure sono doverosi - di sostegno alla popolazione, di creazione dei presupposti affinché il Governo (non fantoccio, ma reale) di Karzai possa avere una forza autogena e capace di dispiegarsi, quando è necessario, in termini di reazione tanto di carattere interno, quanto di carattere oppositorio, se il pericolo viene da fuori dei confini o vicino ai confini. Ci poniamo il problema se le forze che abbiamo mandato debbano svolgere un ruolo militare,

abbiamo avuto il piacere, dal punto di vista della notizia, di ascoltare alcuni rappresentanti di quei gruppi, di quei soggetti che svolgono meritoriamente un ruolo non governativo di sostegno alla popolazione.

una presa di contatto non a livello diplomatico, ma a livello di diplomazia dal basso, che viene ritenuta oggi uno strumento più idoneo di quelli tradizionali. Qualcuno si è scordato di cosa è il ricatto, che cosa è l'estorsione, che cosa è la disparità di condizioni in cui chi è privato della libertà e teme per la vita si trova di fronte ad un soggetto il quale può fare di lui quello che vuole. Si può ritenere che vi sia una legittimazione dal basso verso l'abisso del delitto per consentire un rapporto in cui lo Stato sì prostituisce e si abbatte? Possiamo ritenerlo.

Ma credete voi che sia possibile che un simile avvenimento possa essersi verificato in una situazione nella quale la controparte è diventata addirittura un soggetto con il quale stabilire poi una relazione politica?

tale, divisa tra gli irriducibili, di cui si aspettano i responsi con tremore, ed i riducibili, dai quali si ottiene, nonostante la loro posizione, una acquiescenza.

quello che il senatore Villone ha detto, si possa votare una missione di cui non si è condivisa, né all'inizio, né durante, né ora, la realtà significa trasformare un'opinione legittima e fortemente radicata nella propria coscienza in un atto di acquiescenza politica, invece che di coscienza politica. È un'acquiescenza, perché bisogna consentire che le cose proseguano allo stesso modo, che lo spettacolo continui, che la maggioranza perduri, che vi possa essere, anche con l'aiuto dell'opposizione - è stato detto - una specie di salvacondotto rispetto alle vostre differenze interne.

nella sventura in cui ci capita di vivere, se tutto questo voi lo confondete con una specie di ciambella di salvataggio che stabilisce la prosecuzione, nonostante la vostra incapacità di stare insieme se non convincendo gli irriducibili o convincendo ulteriormente i riducibili, allora mi permetto di dire che forse dovreste riflettere anche su un ultimo punto ultimo punto evidenziato dal nostro ambasciatore: una tensione più alta a Ovest, comprese le vicinanze di Kabul, per allarmi di attentati, mentre i nostri soldati sono ingaggiati (nel senso che sono ingabbiati) con armamenti e con situazioni di autodifesa che corrispondono non alla finalità di un esercito degno di questo nome, ma persino a chi deve svolgere - come la nostra volontà vorrebbe - un compito di salvaguardia della dignità di un Paese e della libertà di un popolo contro chi lo opprime e contro gli assassini tagliagole, con i quali secondo noi non è possibile stabilire alcuna relazione. siamo oggi qui per discutere il rifinanziamento di ventidue missioni militari all'estero: la prima considerazione da fare è che esse sono troppe per le forze di un Paese di media potenza come l'Italia. Tuttavia, fra tutte, due sono le principali missioni: la partecipazione all'ISAF in Afghanistan e all'UNIFIL in Libano. In entrambe manteniamo più o meno la stessa quantità di truppe, sosteniamo all'incirca un'uguale spesa si avvicina anche il numero di Paesi partecipanti che formano il contingente globale dislocato in quelle aree; un abisso politico, però, separa le due missioni.

Abbiamo parlato con quasi tutte le forze politiche del Paese, drammaticamente divise fra di loro; un punto, però, le univa: tessere gli elogi dell'UNIFIL. Il mandato imposto dalla risoluzione 1701 dell'ONU è di essere interposizione fra due avversari; il compito di bloccare una guerra è svolto in modo egregio, la relazione con la popolazione è corretta ed i militari si sforzano di portarle aiuto, soprattutto raccogliendo migliaia di bombe *cluster* di fabbricazione statunitense che i militari israeliani hanno seminato nei campi del Sud dell'antica Fenicia. Il comando sia del capo di tutta l'UNIFIL, il generale di divisione Claudio Graziano, sia del comandante delle truppe italiane, il generale di brigata Paolo Gerometta, mi è parso responsabile, umano ed autorevole, mentre la truppa ben motivata, impegnata ed organizzata. Non ho motivo di credere che le truppe italiane siano differenti in Afghanistan: infatti, appartengono alla stessa scuola; allora, perché considero che esista una distanza immensa fra le due presenze? perché in Libano le truppe sono caschi blu e, in ultima istanza, rispondono al Segretario Generale delle Nazioni Unite; in secondo luogo, perché in Libano i Paesi partecipanti rappresentano un'ampia gamma di culture e collocazioni diversificate nel Pianeta (infatti, vi sono europei, africani ed asiatici; anzi, è da notare una nutrita presenza cinese, qualcosa - fino ad ora - di insolito nelle missioni internazionali); in terzo luogo, perché la risoluzione 1701 è limpida e condivisa (si tratta di un'interposizione fra avversari e della facilitazione di un processo di pace); Libano non è sentita dalla popolazione locale né da altri Paesi del globo come un tentativo di egemonismo da parte di una potenza o di un blocco militare. In Afghanistan, invece, l'offensiva è iniziata come un'invasione da parte degli Stati Uniti all'interno del concetto di «*Enduring Freedom*», cioè della lotta globale contro il terrorismo. Ora, se un'organizzazione criminale come Al Qaeda ha realizzato un attentato mostruoso del tenore di quello alle Torri Gemelle a New York, si doveva attuare un'operazione New York, si doveva attuare un'operazione di polizia, non la mobilitazione di eserciti in metà del mondo (ad esempio, distruggendo l'Iraq, creando prigioni clandestine*,* diffondendo la tortura, massacrando popolazioni e, insieme, minando il diritto internazionale): tutto ciò pesa nella visione mondiale che si ha della missione in Afghanistan. Lì, oltre il 95 per cento delle truppe straniere presenti appartiene alla NATO ed è sotto il comando degli Stati Uniti: è impossibile non sospettare che questa guerra faccia parte di un progetto strategico maggiore (come, ad esempio, l'accerchiamento della Cina o la preparazione di un futuro apocalittico). Le truppe della NATO sono viste dalla popolazione come invasori brutali, che non esistano a devastare montagne, bombardare villaggi e sparare nelle città: ogni giorno si vede lievitare l'odio e crescere la tensione.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, voi tutti ricorderete che nel mese di dicembre del 1979 ebbe inizio l'occupazione militare dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica.

italiani. I miei interlocutori cercarono di motivare la loro decisione adducendo una sorta di loro missione per garantire sicurezza e legalità in quel Paese preda di tremende e sanguinose lacerazioni. In qualche modo, motivarono il loro agire come atto volto a promuovere contemporaneamente progresso civile e sociale. Una volta, forse, avrebbero anche potuto parlare di esportazione dei principi della rivoluzione,

convinzione che soltanto le nostre fossero giuste. Fu un discorso saggio. In conclusione, eravamo concordi nel condannare l'intervento armato compiuto dai sovietici con la pretesa, e nella presunzione, di voler cambiare quella società, in verità volto ad occupare una posizione strategicamente fondamentale a cavallo tra tre continenti: Asia, Africa ed Europa. Oggi, alla stessa stregua, diremmo no all'occupazione militare compiuta dagli americani con la pretesa, e nella presunzione, di esportare con le armi la democrazia.

mentre ora siamo nel 2007. L'intervento servì a cacciare il Governo complice dei terroristi di Bin Laden. Bene: ma sono trascorsi sei anni e l'intervento è divenuto occupazione. ha l'avallo dell'ONU, sì, ma sempre di occupazione, e militare, si tratta. La condizione dell'Afghanistan è rimasta molto grave a causa della mancanza di sicurezza,

non ha accettato di aumentare il numero dei nostri militari, non ha modificato le regole d'ingaggio e sta lavorando per una conferenza di pace seria, tentativo di impegnare gli Stati confinanti, a partire dal Pakistan e dall'Iran; i grandi Paesi che possono essere, e sono, interessati, quali Russia, Cina e India;

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in questo dibattito perché ritengo che gli argomenti

anche di strategia. Una politica estera che, dopo la caduta del Muro di Berlino, ha dato un carattere ulteriore a tutte le iniziative che ci siamo raccontati in questi ultimi anni. Oggi non possiamo negare che, dopo

di politica estera che fa parte del bagaglio sociale, culturale, ma soprattutto politico, di una italianità che, in Europa e nel mondo, si è caratterizzata nel corso degli anni. Ma su questa posizione del Governo

presa d'atto del Governo di non avere una maggioranza, né sulla politica della difesa, né sulla politica estera del nostro Paese, su argomenti strategici che riguardano il futuro non solo dell'Italia, ma delle nuove generazioni di italiani. Abbiamo assistito ad una crisi aperta e chiusa, velocissima, durante la quale i problemi di politica estera non sono stati risolti. Abbiamo visto in Parlamento la riedizione di un Governo, nonostante le dichiarazioni che nulla sarebbe stato come prima se la maggioranza non avesse avuto il consenso in quest'Aula. Invece, nostro malgrado, abbiamo assistito - lo ribadisco - alla ripetizione, alla riedizione di un Governo; abbiamo assistito ad un compattamento su un voto di fiducia di carattere generale. Questo, signor Presidente, signor vice ministro Intini, la dice lunga sulla capacità di tenuta su argomenti importanti, come quelli della politica estera e della difesa, del Governo, che a mio parere è più attento a mantenere posizioni

Ci troviamo di fronte al tentativo rocambolesco da parte del Governo di accomodare, con artifizi, anche dialettici, e documenti più o meno credibili, l'assetto interno di una maggioranza che vede arrivare

Volevo sottolineare questo aspetto perché la dice lunga su quello che sarà il futuro, vice ministro Intini. Ci rendiamo conto delle difficoltà, tant'è vero che in molte occasioni l'UDC ha dato garanzia e disponibilità - e non per il rispetto di equilibri che non vogliamo assolutamente garantire - a non far fare brutta figura al nostro Paese a livello internazionale, agli impegni presi nei fori internazionali, all'adesione al Patto Atlantico e a tutto quello che è stato il codice genetico della nostra caratterizzazione in questi ultimi periodi. Pertanto, quando si parla di terrorismo,

militari, al tentativo di dare un contributo alla lotta contro il terrorismo ci troviamo davanti proposte politiche che non sono quelle di rivedere le regole di ingaggio,

Ascoltavo il senatore Cossutta che giustamente con grande franchezza ha espresso la propria avversità a queste missioni. Ma questo, amici e colleghi senatori, necessita di una conseguente azione politica, occorre votare contro le missioni se crediamo che il voto contrario sia un deterrente. Non bisogna rimanere in maggioranza appoggiando la continuità della politica estera nel nostro Paese. Paese. Rivedere le regole di ingaggio credo sia la conseguente azione di un Governo e di un Parlamento per rispondere a quelle famose minacce che il ministro D'Alema ha denunciato all'opinione pubblica: i nostri soldati sono a rischio. Noi, davanti a questo rischio, cosa facciamo? Siamo partecipi, o meglio non siamo partecipi, del tentativo di liberare il nostro giornalista del

che probabilmente da domani saranno impegnati a sparare contro i nostri militari. Credo che la credibilità di un Governo, ma non solo di quello italiano, si misuri con la grande forza di alcuni Paesi europei di non accettare ricatti di questo tipo che ledono la credibilità di un Paese e che il giorno dopo fanno vedere l'Italia come il ventre molle di una politica europea che, a mio parere, dovrebbe essere forte. Facciamo tutto il possibile, in maniera *bipartisan*, per evitare rapimenti di questo tipo e che i nostri soldati siano oggetto di vessazioni, ma soprattutto non facciamo una politica che indebolisce non solo la nostra politica estera, ma anche l'incolumità dei nostri soldati. Credo che oggi il Governo stia portando avanti una politica che mette in seria discussione

Sul terrorismo non possiamo fare sconti e la Conferenza di pace, proposta alle Nazioni Unite dal Ministro degli esteri, è sicuramente un'iniziativa alla quale guardiamo con attenzione, ma in questo momento pare più il tentativo di acquietare la parte estrema della maggioranza che non un'iniziativa politica di grande respiro. che il segretario del partito di maggioranza della coalizione che sostiene il Governo, l'onorevole Fassino, abbia dichiarato che in quella

di questa leggerezza in politica estera. Siamo preoccupati di come si sta portando avanti la politica nel nostro Paese e soprattutto anche del fatto che le dichiarazioni di questa preoccupazione e di questo sentimento vengono scambiate per turbolenze domestiche. Questi sono sentimenti degli italiani. Dobbiamo difendere la credibilità del nostro Paese, dobbiamo dare forza alla continuità. Per questa ragione voteremo a favore del provvedimento, per la continuità della politica estera del nostro Paese. Soprattutto, dobbiamo mettere in campo - e concludo

La mia opinione a favore del decreto si fonda sul fatto che questo provvedimento rappresenta un momento importante dello sviluppo della politica estera del nostro Governo. In primo luogo, l'attenzione va ai grandi problemi dello scacchiere del Medio Oriente e di quello asiatico.

Forse occorrerà nei prossimi mesi valutare come consolidare i processi politici che possono condurre ad una pace duratura, a partire dal sostegno al dialogo tra Israele e il nuovo Governo di Palestina. Qui si pone un punto di grande importanza e delicatezza, non meno importante che nelle altre missioni. Oltre alle altre missioni sullo scacchiere internazionale, voglio solo ricordare in maniera veloce ma importante quella in Kosovo, su cui, però, sarebbe utile ritornare, riservando una discussione in relazione alla nuova realtà che dobbiamo affrontare in

Noi riconfermiamo la nostra presenza in quel Paese sulla base di una considerazione politica oggettiva (lo dico io che ho avuto dubbi, critiche e anche contrarietà a questa presenza): solo con la guerra non si risolve il problema dell'Afghanistan. La guerra perenne, che ormai dura da sei anni, non solo non è una soluzione, ma rischia di ritorcersi, e si ritorce, contro chi la predica. Il rischio della guerra perenne potrebbe essere una sorta di ecatombe, come sta succedendo in Iraq. L'esportazione della democrazia con sessanta morti al giorno non avviene. La nostra missione, quindi, ha il carattere di chi vuole mantenere il proprio ruolo militare rispetto agli altri Paesi. Accentuare il ruolo militare significa non solo comprendere ciò che viene avanti, ma anche intervenire più efficacemente sulle questioni della cooperazione, per affrontare i problemi di ogni giorno delle popolazioni civili. I contatti che ognuno di noi con la società civile afghana ci fanno comprendere questo. Anzi, vi è stanchezza nei confronti della presenza degli stranieri. Lo ha già ricordato il senatore Cossutta, ma anche il senatore Villone.

Questo deve insegnarci qualcosa. Oggi il problema è prettamente politico. La Conferenza internazionale non è un'invenzione, né un'esigenza astratta

Quindi, l'importante è entrare in una fase che impedisca, appunto, l'«irachizzazione» dell'Afghanistan, cioè una situazione senza ritorno.

*(UDC)*. Signor Presidente, l'UDC è solidale con i nostri soldati che in diversi Paesi del mondo oggi difendono la pace e la possibilità di un avvenire migliore per i popoli tra i quali sono impegnati. Siamo fieri di ciò che stiamo facendo nei Balcani. Sono stato nel Kosovo settentrionale e ho visitato i monasteri serbi, dove i monaci mi hanno ringraziato, dichiarandomi che se non ci fossero stati i soldati italiani, sarebbero già morti o dovuti fuggire. Siamo convinti che non sia possibile rinunciare all'uso della forza al servizio dei diritti dell'uomo e sappiamo che i pacifici non coincidono necessariamente con i pacifisti. Anch'io ho qualche memoria, senatore Cossutta, e ricordo i cortei dei pacifisti, quelli che manifestavano contro l'installazione dei missili in Germania. Poi abbiamo scoperto che erano pagati dai servizi segreti della DDR. Diffido di quel tipo di pacifismo. Siamo preoccupati e orgogliosi al contempo. Siamo preoccupati per la situazione in Libano, perché siamo lì per un missione specifica che è quella di appoggiare l'esercito libanese che deve disarmare Hezbollah.

di una guerra nella quale non sappiamo bene quale sia il nostro compito. Seguiamo con attenzione quella realtà. Chiediamo un'iniziativa più forte, perché la missione originale venga ripristinata. Oggi ci pare alquanto nebulosa. Siamo in Afghanistan per un decisione del Governo Berlusconi presa nel quadro della NATO e con l'avallo delle Nazioni Unite. Ma perché siamo in Afghanistan? L'Unione Sovietica andò in Afghanistan con un colpo di stato, per sottomettere un popolo che non voleva essere sottomesso. Noi non siamo andati in Afghanistan per esportare la democrazia; vi siamo andati per distruggere le basi da cui era partito l'attacco contro le torri gemelle di New York. Questa è la vera questione, che vedo poco ricordata in questa Aula: c'è o non c'è una guerra contro il terrorismo? C'è o non c'è la minaccia di un terrorismo internazionale, che occupa alcuni Stati e ne fa proprie basi di partenza e che domani potrebbe essere dotato di armi nucleari? Esiste o non esiste il problema di evitare che le armi nucleari vadano nelle mani di governi che potrebbero utilizzarle per fini di terrorismo internazionale? Esiste o non esiste il problema di un attacco violento, che mira a prendere in mano l'intero Medio Oriente? Vedete, quello che succede in Afghanistan ha effetti immediati su quello che succede in tutto il Medio Oriente. C'è la volontà di scuotere il prestigio dei governi moderati davanti alle loro popolazioni; c'è un progetto lucido per acquisire il controllo dell'intera area mediorientale, per ricostruire il califfato e condurlo alla guerra santa contro l'Occidente. Queste sono le ragioni per le quali oggi noi siamo in Afghanistan. Se non abbiamo chiare le ragioni, non abbiamo chiaro neanche perché ci stiamo; diventa allora difficile sostenere la presenza dei nostri soldati. C'è o non c'è un pericolo? Se non c'è un pericolo, devono tornare a casa; se c'è un pericolo, sono in Afghanistan per tenere quel pericolo lontano dalle nostre case. E sono in Afghanistan con una missione che è una missione militare. Le popolazioni locali si aspettano, certo, di ricevere aiuto e sostegno economico, civile, sociale; si aspettano che i nostri soldati sappiano costruire le strade o addestrare la polizia. Ma, prima di tutto, si aspettano che i nostri soldati sappiano usare le armi per difenderle dai loro massacratori. Vi ricordate Srebrenica? Truppe di un esercito alleato, prive di direttive adeguate, prive di armamento adeguato, lasciarono che sotto i loro occhi fossero massacrate 7.000 persone, macchiando la bandiera del loro Paese di una vergogna indimenticabile. Lì vicino, il generale Morillon schierò i soldati francesi a difesa delle popolazioni affidate alle sue cure e dichiarò in modo credibile che avrebbe aperto il fuoco; lì, allora, il massacro non ebbe luogo. Questo è il problema. Avete letto in che modo hanno sgozzato quel povero ragazzo che accompagnava il nostro giornalista? Ecco, questo è il problema. Siamo in grado di garantire questa protezione? Perché siamo lì per garantire questa protezione; questa è la finalità prima, tutto il resto la accompagna. Per svolgere questa missione i soldati devono essere adeguatamente addestrati, avere supporto logistico e regole d'ingaggio adeguate alla loro missione. È difficile per noi capire per quale motivo il Governo possa dire di no ad una mozione, come quella della Lega, in cui gli si chiede semplicemente di garantire che i soldati possano svolgere la loro missione. O forse c'è la preoccupazione di chiedere i nostri voti e di blindare contemporaneamente la propria maggioranza? Sono due finalità contraddittorie, le quali non possono essere perseguite contemporaneamente. Noi chiediamo un miglioramento dell'equipaggiamento pesante, chiediamo regole d'ingaggio adeguate, chiediamo un'integrazione più forte con le truppe dei Paesi alleati. Non è pensabile che noi ci riserviamo di non andare in aiuto loro, quando sono attaccati, e poi pensiamo che loro vengano volentieri in aiuto nostro, quando fossimo attaccati noi. Questo ci sembra non sufficientemente chiaro. Siamo preoccupati per lo smantellamento dei servizi segreti, conseguente alla gestione malaccorta dei casi Abu Omar e Calipari. Chi si fida oggi di servizi segreti che possono essere obbligati a manifestare i nomi dei loro informatori o le procedure che hanno seguito nella soluzione di un problema? soluzione di un problema? Chi telefona ai servizi segreti italiani, sapendo che la sua conversazione potrebbe essere ascoltata dalla magistratura? E non diteci che c'è il segreto istruttorio, per carità di patria, non parliamo di questo problema! Questo è preoccupante, perché queste guerre si fanno con i servizi segreti. Sono guerre lunghe, sono guerre difficili, sono guerre che chiedono grande determinazioni. La Conferenza di pace può essere utile, ma non facciamoci illusioni: la Conferenza di pace vera ci sarà quando i talebani saranno stati debellati. Si poteva fare una conferenza di pace con la Germania nazista nel 1942, nel 1943 o nel 1944? Ecco, domandiamoci i talebani sono disposti a sedere in una Conferenza di pace senza chiedere che vengano consegnate quelle povere popolazioni nelle loro mani perché le possano massacrare a loro piacimento? Perché, se non sono disponibili a sedersi, la Conferenza può essere sempre utile per avere un aiuto da tutti i Paesi intorno per tagliargli i rifornimenti e ripristinare condizioni migliori ma certamente non sarà decisiva; diventa come un sigaro che non si nega a nessuno, tanto più quando un Governo come quello italiano ne ha assolutamente bisogno per dare una qualche impressione di accoglienza delle tesi di una parte della sua maggioranza. Siamo preoccupati per la debolezza del sostegno politico che questo Governo è in grado di dare ai nostri soldati. Se passa l'idea che siamo l'anello debole della catena tutti gli attacchi si concentreranno contro i soldati italiani; e non pensate che siamo in un'area tranquilla, potrebbe rapidamente diventare un'area di grande impegno militare. Per queste ragioni ragioni l'UDC darà il suo voto a sostegno dei nostri soldati. Ci aspettiamo però che i nostri voti si aggiungano e non si sostituiscano a quelli della maggioranza. Se così fosse il Governo avrebbe il dovere morale e politico di dimettersi. Se non lo facesse sarebbe questa una grave violazione delle regole di una democrazia matura. Il Governo si metterebbe in un certo senso fuori legge e non potrebbe certo lamentarsi se poi in altra occasione queste regole non fossero osservate da parte delle opposizioni. Il Governo ha garantito al Capo dello Stato di avere una maggioranza per governare, in particolare la politica estera del Paese. Se nei fatti risultasse che questa non esiste allora la fiducia che la maggioranza ha ottenuto in quest'Aula risulterebbe essere una pantomima, che offende sia il Capo dello Stato che la nazione italiana. Sarebbe una fiducia per durare e occupare il potere, non per governare. Un Governo che governasse con una simile fiducia non potrebbe garantire ai nostri soldati quel supporto cui hanno diritto e la soluzione potrebbe essere solo una: le sue dimissioni. Sarebbe anche un atto umanitario verso gran parte dell'opposizione, che vota contro la propria coscienza soltanto per mantenere in piedi un potere nel quale non può credere.

La vita è tutta una lezione. Per esempio, la seduta di oggi e i discorsi dell'opposizione che ho ascoltato fino ad ora mi hanno svelato che non di guerra, non di terrorismo, non di talebani, non di sostegno all'America, non di sangue, non di pericolo, non di morte, non di incursioni si sta sta parlando; si sta parlando del vero pericolo dell'umanità, che è Romano Prodi e il suo Governo. E si sta parlando, come ha fatto un momento fa il senatore Buttiglione per volte, di dimissioni o di necessità di dimissioni, perché è il punto fondamentale. Bisogna che il Governo Prodi se ne vada:, è l'ordine che è stato dato

che il problema è quello. L'altra cosa che ho imparato è che i fedeli seguaci del capotribù non hanno alcuna difficoltà ad essere in perfetto contrasto con se stessi e ci dicono delle cose che sono l'opposto esatto di ciò che ci hanno detto quando erano al Governo. Quando erano al Governo ci hanno detto che si trattava di missioni di pace e hanno tuonato. Ricordo quando ero direttore de «l'Unità» e mi permettevo di dire: come può essere missione di pace quella di un contingente di soldati italiani messi al servizio di due armate in guerra? Venivo investito da vere e proprie maledizioni, sia nel nei *talk show* e nelle televisioni controllate dal gruppo di cui stiamo parlando, cioè tutte, sia dai giornali, vuoi quelli di proprietà, vuoi quelli in cui è più prudente per un giornalista italiano mettersi dalla parte di un grande editore che mettersi contro.

noi avevamo detto: accidenti, siamo sicuri che alla luce dell'articolo 11 della Costituzione si possa impegnare l'Italia in un'azione di guerra? Questa mattina, nella giornata di oggi, e da quando stiamo discutendo del rinnovo della missione, pur di far cadere il Governo Prodi, l'articolo 11 della Costituzione non esiste più. non c'è più alcuna preoccupazione tanto che sostenete che, va benissimo, questa è guerra. In secondo luogo abbiamo sentito dire che i nostri soldati non sono militarmente dotati di tutte le strutture che servirebbero loro per difendersi. Benissimo,

di quello che succedeva ed è successo agli ostaggi che avete liberato. Ci siamo compiaciuti, lo ha detto questa mattina il capogruppo dell'Ulivo, siamo stati molto felici che siano stati liberati e che siano tornati vivi. Ci siamo compiaciuti, ma non abbiamo potuto sapere nulla perché mai nulla è stato detto o rivelato.

quando con una Conferenza di pace si toglierà ai talebani quel territorio di rifugio e di compensazione continua che è il Pakistan, dal quale vengono continuamente riforniti, godendo di quella ripresa di possibilità che li conduce ad una guerra infinita. Ecco, la guerra infinita non è nella prospettiva della nuova democrazia americana, non è quello di cui sta parlando la Commissione esteri del Senato americano, non è quella di cui parla sul «New York Times» di oggi, invocando

Romano Prodi, che volete abbattere in tutti i modi, trascurando completamente il Mullah Omar e tutti i personaggi del terrorismo, che vi stanno a cuore solo secondariamente, perché il compito più importante è quello di far tacere e di far cadere l'attuale Governo. Bene, può anche darsi che esso non cada: in quel caso continueremo a scambiarci opinioni su come fare la pace in Afghanistan e nel resto mondo Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il tempo oggi a mia disposizione è troppo breve per esaminare la questione Afghanistan sotto tutti i diversi delicati profili che presenta. Limiterò pertanto il mio intervento ai due punti che ritengo più urgenti. In primo luogo, chi parla è seriamente preoccupato per le condizioni nelle quali si trovano ad operare i nostri militari impegnati sul fronte afghano. È noto che, con la primavera imminente, si annuncia la tanto attesa offensiva talebana, della quale il rapimento del giornalista Mastrogiacomo è stato solo un'avvisaglia. Come si stanno preparando i nostri soldati? Tutti gli osservatori e i giornalisti rientrati dal teatro di operazioni del nostro contingente denunciano la fragilità e l'inadeguatezza del dispositivo difensivo a loro disposizione. Mentre gli altri contingenti, compreso quello spagnolo, che opera nello stesso scacchiere di Sud-Est, hanno dotato di armamento pesante i loro soldati ed hanno inviato in Afghanistan blindati ed artiglieria, i nostri Comandi, per espresse istruzioni impartite da Roma, non prendono contromisure e mantengono un dispositivo leggerissimo, dotati al massimo di mitragliatrici. Non ci sono cannoni, né mortai, né veicoli corazzati, né elicotteri a prova di proiettile. Il mezzo più potente a disposizione sono le autoblindo «Puma», che non hanno nemmeno le torrette per proteggere i mitraglieri, obbligati a fare da bersaglio per i cecchini, né corazzature aggiuntive contro i micidiali ordigni esplosivi in dotazione ai terroristi talebani, mentre i più potenti blindati «Centauro» sono schierati in Libano, perché magari, secondo alcuni esponenti della maggioranza, devono fronteggiare l'esercito israeliano. Come chi parla ha già denunciato in una recente interrogazione, rimasta come al solito senza risposta, il nostro contingente, privo com'è di appoggio politico da parte del proprio Governo e di solidarietà militare, è esposto addirittura alle ironie della stampa afghana, che proprio qualche giorno fa ha riprodotto una vignetta inglese risalente alla seconda guerra mondiale, secondo cui «i carri armati italiani hanno cinque marce, una avanti e quattro indietro». Purtroppo la storia si sta ripetendo. La situazione venutasi a creare in Afghanistan mi ricorda infatti, per certi versi, quella descritta da Giulio Bedeschi in «Centomila gavette di ghiaccio» o da Mario Rigoni Stern ne «Il sergente nella neve», quando nel secondo conflitto mondiale i nostri alpini vennero mandati dal regime fascista a combattere e morire in Russia, con temperature glaciali ed equipaggiamenti del tutto inadeguati per quel teatro di operazioni. Ironia della sorte, anche oggi in Afghanistan sono schierati dei reparti alpini. Voglia Iddio che, nelle prossime settimane, nessuno dei nostri militari abbia a pagare con il sacrificio personale questa irresponsabile scelta del nostro Governo. Non vi è dubbio che, fino ad oggi, la nostra missione ha svolto un ruolo essenzialmente umanitario, ma se, come ha recentemente detto il sottosegretario per la difesa Forcieri, «anche se non cerchiamo guai, i guai cercheranno noi», è necessario garantire al meglio la vita e la sicurezza dei nostri soldati. Guarda caso, proprio ieri alcuni militari del nostro contingente sono stati oggetto di un attacco terroristico e uno di loro è rimasto anche leggermente ferito. Nelle stesse ore, il ministro D'Alema a New York ha dichiarato: «La guerriglia sta arrivando anche a Herat e non credo che le truppe italiane siano in una buona situazione. Affronteremo momenti difficili». Questo ha detto proprio ieri, senatore Colombo, il Ministro degli affari esteri! Quindi, se queste sono le condizioni sul terreno e se lo stesso Governo è consapevole della criticità della situazione venutasi a creare nel teatro di operazioni, è necessario ed urgente che le nostre truppe siamo messe quantomeno in condizione di difendersi con la massima efficacia, di fronte all'aggressione nemica. È per questo che condivido in pieno l'ordine del giorno che il presidente del mio gruppo, senatore Schifani, ha presentato come contributo a questo dibattito, con l'invito al Governo ad impegnarsi per l'invio immediato in Afghanistan - ad uso difensivo, beninteso - del più efficace equipaggiamento e dei migliori sistemi d'arma di cui è dotato il nostro esercito, per fornire un deterrente credibile e un'adeguata capacità di reazione. Su questo punto, credo, il Senato non dovrà dividersi, perché siamo chiamati a garantire la sicurezza dei nostri militari, senza peraltro modificarne il quadro generale d'intervento. Sarebbe invero molto grave, anzi sarebbe un errore madornale, se la maggioranza respingesse tale ordine del giorno. Di quale insopportabile responsabilità si renderebbe complice quest'Aula? Cosa dovrebbero pensare i nostri militari impegnati in Afghanistan? E cosa potrebbe pensare il Paese? Che il Parlamento non ritiene necessario tutelare al massimo le vite dei militari impegnati all'estero? Le conseguenze per la tenuta della missione sarebbero davvero devastanti. secondo luogo, e concludo, siamo tutti soddisfatti e tranquillizzati per la liberazione del giornalista Mastrogiacomo. Ma ci rimane un dubbio. Perché, dopo aver ottenuto dal Governo afghano il rilascio il rilascio di ben cinque capi talebani, chi ha condotto la trattativa non si è preoccupato di ottenere, insieme a quella di Mastrogiacomo, anche la liberazione dell'interprete afghano Ajmal Nashkbandi, di cui invece non si hanno notizie e che pare sia ancora nelle mani dei terroristi? Mi pare di capire che in questo caso c'era un ostaggio di serie A,

*(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a discutere su un argomento di straordinaria importanza per la politica estera del nostro Paese e vitale per la temporanea sopravvivenza del Governo Prodi. Infatti, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene, com'è noto, disposizioni volte a prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane alle missioni internazionali di aiuto umanitario.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 Credo che questo disegno di legge, nel momento in cui si prefigge di reiterare gli aiuti umanitari e gli stanziamenti di cooperazione allo sviluppo nei confronti di tale Paese, presenti, però, un'incongruenza di fondo, una contraddizione intrinseca che mina l'intera architettura della politica estera italiana. Limito, per motivi di tempo, la mia analisi a due scenari: l'Afghanistan e il Libano. L'intervento in Afghanistan, come tutti sanno, fu deciso dalla quasi unanimità della comunità internazionale, in seguito alla risoluzione n. 1386 del 2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che istituì la forza di intervento ISAF. Da allora si è proceduto ad una progressiva stabilizzazione del Paese che, però, negli ultimi anni ha registrato una risorgenza dell'attività terroristica dei gruppi talebani, notoriamente legati ad Al Qaeda, che ha posto le Nazioni Unite e, in particolare, le forze NATO operanti sul terreno, di fronte all'esigenza di contrastare militarmente tale recrudescenza. Di fronte a tale situazione, la posizione del Governo italiano permane evasiva e ambigua, per non dire del tutto latitante. Nel disegno di legge al nostro esame si prevedono misure, sicuramente opportune, di aiuto umanitario per le popolazioni afghane, ma non si dice nulla circa la posizione che le nostre truppe devono tenere sul campo. Ciò è grave soprattutto alla luce del fatto fondamentale che il contingente italiano è schierato e integrato con i nostri alleati dell'Alleanza atlantica, la quale ha esplicitamente richiesto a tutti i Paesi coinvolti di incrementare l'operatività delle unità militari *combat ready*. A questo proposito, chiedo al Governo quali saranno le regole di ingaggio cui i nostri soldati dovranno adeguarsi nei prossimi mesi in questo martoriato Paese. È possibile continuare a perseguire una politica ambivalente, in cui noi ci occupiamo solo di aiuto umanitario, o auspichiamo conferenze di pace con i terroristi, mentre i nostri alleati accrescono le forze militari che contrastano la rinascita dei talebani? Non ritiene l'attuale maggioranza che tale comportamento sia altamente nocivo per l'appartenenza stessa ad un'Alleanza, quella transatlantica, che costituisce l'alfa e l'omega della nostra politica estera? Ricordo che l'Italia, dalla nascita della Repubblica, si è sempre basata su tre linee direttrici cruciali di politica internazionale: l'Alleanza militare della NATO, l'integrazione comunitaria e la cooperazione mediterranea. Con l'attuale comportamento in Afghanistan e gli avvenimenti di queste ultime ore, noi stiamo, a mio avviso, mettendo a repentaglio uno degli assi portanti della nostra tradizionale proiezione diplomatica, perché mostriamo chiaramente di non voler condividere l'orientamento di un'Alleanza che ci chiede non solo l'assistenza finanziaria e umanitaria, ma anche di combattere contro il nemico comune al quale, al contrario, siamo noi stessi, purtroppo, a fornire ulteriori mezzi per combatterci. La stessa aporia è data rilevare nell'approccio dell'attuale Governo sul Libano. Qui, ancora una volta con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la 1701 dell'agosto 2006, si è proceduto a dispiegare un contingente militare di interposizione, in cui risalta la cospicua componente italiana, tant'è che è guidato da un generale italiano.

I maggiori analisti diplomatici riconoscono che l'allentamento della tensione in questo Paese sarò possibile solo quando verranno smantellati tali gruppi armati, solo quando verrà restituita a questo Paese la sua esplicita e completa sovranità, solo quando non ci sarà più uno Stato nello Stato come è attualmente. Anche a questo riguardo, l'attività del Governo italiano si è contraddistinta per la sua unilateralità: si è preferito invocare il solo ritiro delle truppe di Israele, quando invece sarebbe stato opportuno richiedere, insieme a tale ritiro, anche il disarmo di Hezbollah e di tutte le altre milizie non inquadrate nell'esercito ufficiale del legittimo Governo libanese. Ancora una volta, dunque, la nostra politica estera ha fatto registrare una caratteristica intrinseca di ambiguità e, soprattutto, di divaricazione con gli interessi primari e prevalenti del nostro Paese, che sono quelli di essere accanto ai Paesi democratici, di sviluppare efficaci e realistiche azioni di pace e di salvaguardare i principi basilari su cui riposano le nostre società occidentali. che in Afghanistan ne risulta gravemente minata la credibilità dell'Italia verso i nostri interlocutori europei e verso il *partner* americano. Ma non lo dico solo io: come ha rilevato oggi Piero Ostellino sul «Corriere della Sera», la politica estera guidata dai movimenti e da Emergency esautora il ruolo dello Stato italiano, svilisce e nullifica la nostra diplomazia. Noi esprimiamo la nostra più viva solidarietà a tutte le Forze armate e di polizia che operano in nome della libertà e della democrazia con grande competenza e con spirito di sacrificio non solo nei Paesi interessati dal decreto-legge oggi in esame ma anche nelle altre parti del mondo.

Il disegno di legge su cui oggi ci troviamo a discutere rappresenta la concreta risposta del nostro Paese alla sfida per il raggiungimento di pace, democrazia e benessere che l'Italia si è imposta di perseguire attraverso le sue missioni umanitarie in molte zone del mondo, sempre - ci tengo a ricordarlo - nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei princìpi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. E leggendo il documento in questione non si può non notare il profondo e sentito interesse per il raggiungimento degli importanti obiettivi in quei territori che oggi sono scenario di tensioni e conflitti, e la volontà di andare avanti e portare a conclusione, nel migliore dei modi possibile, delle missioni che non dimenticano i civili, la parte più debole e più colpita di Paesi vessati da conflitti e povertà, ma che hanno come punto centrale proprio la collaborazione con le popolazioni locali, oltre a una crescente attenzione agli aspetti della cooperazione civile. Il confronto avviato nelle Commissioni dimostra l'impegno forte e costante, delle diverse parti politiche, nel perseguire e raggiungere gli obiettivi che l'Italia non può mancare nel difficile contesto internazionale. Le due novità rispetto ai precedenti provvedimenti di proroga sono la fine della missione militare in Iraq, ma non dell'impegno di cooperazione civile in quel territorio, e la prima proroga del finanziamento della missione UNIFIL in Libano, l'impegno più rilevante tra le missioni internazionali del nostro Paese. A tale proposito, vorrei ricordare e ringraziare tutti i militari italiani che operano in tutte quelle zone colpite dai conflitti, portando sollievo e sostegno alle popolazioni civili coinvolte. Un impegno riconosciuto dai nostri alleati, apprezzato in ambito internazionale e guardato con riconoscenza dalle stesse popolazioni locali. Un impegno che - non dimentichiamolo - svolgiamo nell'ambito di un quadro più vasto di collaborazione responsabile con i nostri alleati. E proprio in virtù di questo rafforzamento del multilateralismo in politica estera e del rilancio del ruolo centrale dell'ONU, l'Italia non può sottrarsi in questo momento alla sua funzione sullo scenario internazionale: questo, infatti, significherebbe venir meno agli impegni assunti dal nostro Paese con le Nazioni Unite, con la NATO e con l'Unione Europea. Vorrebbe dire, inoltre, rinunciare al processo di costruzione europea e, ancor più grave, perdere quello slancio contro la povertà e il sottosviluppo nel mondo. Anche perché, per quanto la discussione verta prevalentemente sul tema dell'Afghanistan, il disegno di legge propone di rifinanziare altre importanti missioni in Paesi quali il Libano e il Sudan, Paesi che chiedono aiuto e attenzione da parte della comunità internazionale e che hanno coinvolto, come in Afghanistan, un impegno comune delle forze multinazionali. Signor Presidente,voglio soffermarmi brevemente sul Sudan, del quale si è parlato poco nel corso di questo dibattito. È un Paese che ho visitato più volte e che conosco molto bene. Ho vissuto in Eritrea, quindi ai confini con il Sudan che

regione occidentale situata nel deserto del Sahara, segnata da anni dalla violenza e dal terrore. Ho letto

stupri generalizzati e rapimenti». Ma il documento, signor Presidente, è duro anche con la comunità internazionale, il cui comportamento davanti alla tragedia viene definito dall'ONU «patetico» e alla quale viene chiesto di agire immediatamente per fermare la carneficina in atto

Signor Presidente, onorevoli colleghi, scriveva Sigmund Freud che l'inclinazione degli esseri umani all'abitudine è, insieme, la loro forza e la loro debolezza: resistono a tutto e, contemporaneamente, si abituano all'orrore, alla rassegnazione, alla guerra. Anche dalla guerra, dunque, possiamo proteggerci con il manto dell'assuefazione e, mentre i nostri cacciabombardieri distruggono Belgrado e la Zastava, disseminano l'uranio impoverito sulla terra, sui fiumi e sulle popolazioni della Jugoslavia, mentre i nostri soldati combattono, muoiono e uccidono per una guerra americana in Iraq e in Afghanistan, possiamo continuare cristianamente a vivere con il cuore sereno e ad evocare la pace. Siamo un Paese in guerra, ormai da molti anni e con diversi fronti aperti; ma l'abitudine ce lo fa dimenticare. Ma un Paese in guerra, produce storicamente e necessariamente due effetti tra loro speculari: da una parte, la rimozione, la censura e persino la menzogna organizzata rispetto ai motivi reali della guerra; dall'altra, la militarizzazione interna allo stesso Paese in guerra: il fronte esterno e quello interno, entrambi da presidiare con la medesima durezza e intensità. Accade così anche oggi in Italia: dopo sei anni dall'attacco americano contro l'Afghanistan, quasi nessuno ne ricorda più il motivo scatenante proclamato, ossia la cattura di Bin Laden. Ma poiché non si può invadere un Paese, bombardarlo per sei lunghi anni, distruggerlo in lungo e in largo, ridurre un popolo alla fame e ammazzare 80 mila persone, di cui l'ottanta per cento civili, solo per catturare un uomo, la cultura dominante ha dovuto diffondere - rimuovendo il primo - un nuovo messaggio, più realistico: non bombardiamo per catturare Bin Laden, ma contro i talebani. Sono dunque i talebani - già grandi amici degli USA - il motivo reale della guerra? Nulla è tanto ballerino quanto i princìpi dell'imperialismo. Era Benedetto Croce, alla fine del secondo dopoguerra, a chiedere ai laburisti inglesi di non appoggiare più il fascismo spagnolo, dopo la caduta di Hitler; ed erano i laburisti a rispondergli, per non entrare in rotta con il generale Franco, che si doveva rispettare ovunque, sempre ed anche con sofferenza, il principio sacro dell'autodeterminazione dei popoli e dei Governi; gli stessi laburisti, non solo inglesi, che oggi, al servizio degli USA, sostengono l'intervento militare in Afghanistan. Ma la verità sull'Afghanistan, scientemente censurata, è tutta da un'altra parte. La verità è che il progetto di controllo militare dell'Afghanistan lo si trova teorizzato nelle carte del Pentagono ben prima dell'11 settembre e che tale controllo per la Casa Bianca è parte preponderante e teorizzata del disegno generale di guerra infinita e permanente, dell'estensione della NATO nel cuore dell'Asia, ai confini di quell'Iran da normalizzare militarmente, del Pakistan e, soprattutto, della Cina, ormai primo e strategico avversario degli USA. La verità è che nell'agosto del 2003 la missione ISAF è passata sotto il comando NATO: modo otto le basi NATO costruite - o in costruzione - in Afghanistan e dovrebbero diventare circa venti. Per organizzare tanta capacità di fuoco e controllo egemonico in quell'area strategica, gli USA possono agevolmente mettere nel bilancio di guerra il genocidio del popolo afghano e centinaia, anche migliaia di vittime tra la coalizione occupante. Ma oltre che di costruire una falsa coscienza di massa, un Paese in guerra ha bisogno di aprire e di controllare anche un fronte interno, militarizzando la società, la politica, i partiti. Che cos'altro è, se non una forma di militarizzazione, questo coro filoamericano, questa voce mediatica pressoché univoca, volta a sorreggere e ampliare l'intervento in Afghanistan? Che cos'è questa gabbia di ferro montata attorno al movimento per la pace, questo impressionante tentativo di demonizzare il dissenso sociale e politico, questo pericoloso intento, volto a far abbassare la testa ai deputati e ai senatori? E ancora, che cos'è, se non un vero e proprio trasferimento interno del fronte militare, la minaccia e la pratica dell'emarginazione, dell'espulsione dei dissidenti e dei pacifisti dai loro partiti? Noi non possiamo tradire il nostro popolo, la nostra classe sociale di riferimento, questo è il punto centrale. Ci hanno dato il loro voto per cambiare, per avere il coraggio di essere, almeno un po', autonomi dagli USA, dalla NATO, dal Vaticano, da Confindustria, dai padroni del vapore e dall'Europa di Maastricht. Se deludiamo di nuovo le speranze della nostra gente, allora sì che apriamo le porte al ritorno delle destre. Ci dicono: attenzione alle destre; e hanno ragione, perché siamo di fronte ad una delle più populiste e pericolose destre d'Europa. A questa destra viene voglia di dire, come si faceva un tempo: «*No pasaran*», non passerete, non tornerete al Governo con il mio voto sbagliato. Io mi sento così parte della classe operaia, del suo spirito e della sua materialità ma, contemporaneamente, vorrei dire all'intera sinistra e alla mia coalizione: consegnatelo voi il Governo alle destre con politiche sbagliate, che ci allontanano dal nostro popolo. Bisogna cambiare. Dall'Afghanistan occorre ritirarsi. Dalle politiche di guerra degli USA e della NATO bisogna liberarsi. Da un papato che metterebbe di nuovo al rogo Giordano Bruno occorre emanciparsi. Bisogna frenare questo imponente e pericoloso processo di militarizzazione e dedicarsi molto di più ai salari, alle pensioni, alla ricostruzione di uno Stato sociale, ai diritti civili e di libertà. Sono sempre più contrario alla guerra in Afghanistan ma voterò, per questa volta ancora, le indicazioni del mio partito per non favorire le destre, per non provocare uno spostamento centrista e per non essere emarginato ed espulso dalla battaglia politica futura. Non darò un voto sbagliato, ma chiedo al Governo Prodi di non farmi sbagliare votandolo.

che non disarticolano ma uniscono. Vorrei soffermarmi su alcune obiezioni avanzate dai colleghi della destra a proposito dell'Afghanistan facendo alcune considerazioni sull'andamento della situazione in quel Paese. Schematicamente, la destra si dichiara d'accordo su tutte le missioni militari, ma lamenta che non siamo abbastanza muscolari e all'altezza della situazione, nonostante il Capo di stato maggiore della difesa abbia affermato che i nostri militari sono equipaggiati «al meglio» e che non hanno nulla da invidiare

della responsabilità dell'attuale irachizzazione del Paese e delle prospettive di uscita o di risoluzione da questo disastro. Accanto ad innegabili, ma parziali, dati positivi (li riconosciamo tutti e li diciamo: la ripresa della scolarizzazione, soprattutto per le bambine, un lento avvio del processo di ricostruzione, la poco più che simbolica, ma importante, costruzione di istituzioni democratiche e di un esercito nazionale), permangono elementi di forte preoccupazione (la mancanza di sicurezza, innanzitutto, ma anche la forte ripresa del narcotraffico, il dilagare della corruzione, l'aumento dei bombardamenti a Sud-Ovest), che rendano sempre più drammatiche le condizioni di vita quotidiane. Sulla materialità di questa situazione l'intervento militare è inefficace, non conquista cuori e menti, mentre è proprio sulla delusione e sul malcontento popolare che i talebani possono fare breccia. Detto tra parentesi, il Governatore della confinante provincia pachistana del Belucistan sostiene l'esistenza di un rischio che la guerra dei talebani diventi una guerra di tutto il popolo. Ma non lo si può sterminare tutto! Questa situazione, già critica e che solo nello scorso anno ha causato 4.000 morti (di cui la maggioranza, - lo sottolineo - civili) in scontri e attentati, si è aggravata. Di fronte a questa sempre più drammatica situazione del Paese, qual è l'ipotesi della destra? Armiamoci di più e sterminiamo i talebani! Io non condivido tale soluzione e non per una questione di impegno numerico, come spiegato benissimo stamattina dal senatore Tonini, in riferimento alle ingenti forze degli Stati Uniti in Iraq e della fu Armata Rossa in Afghanistan. Non sono d'accordo su una soluzione muscolare e violenta, anche perché inefficace, controproducente rispetto ad un Paese che ha soprattutto bisogno di essere pacificato attraverso un impegno politico, civile ed economico. Le ragioni urlate dalla destra contro le dichiarazioni di Piero Fassino, favorevole alla partecipazione anche dei talebani alla conferenza di pace sull'Afghanistan, cosa che avevamo chiesto in un ordine del giorno qui al Senato a luglio, a luglio, nascondono la voglia dell'attuale opposizione di sottrarsi in quest'Aula ad un voto favorevole alle missioni internazionali, intento tutto politico e strumentale, volto all'indebolimento del Governo. È sotto gli occhi di tutti che l'uso della forza militare non ha prodotto la stabilizzazione nel Paese. Occorrono politica, trattative, dialogo, diplomazia, ma anche conoscenza, *intelligence*, dissuasione.

che vedeva come merce di scambio la consegna di capi di Al Qaeda contro la fine dei bombardamenti dei campi di addestramento. Forse se (ma la storia non si fa con i «se»)

i quali tutti, indipendentemente dal partito che votano (mi riferisco a quelli di questa parte), non vogliono assolutamente, neppure uno, mai,

Naturalmente, se fosse proposta e riscritta in modo tutt'affatto differente, la situazione sarebbe diversamente affrontabile, ma poiché questa è la realtà, credo di essere interprete di una larghissima,

e che noi ci sforziamo di rappresentare, possibilmente di più e meglio di quanto non cerchiamo di rappresentare le gerarchie di partito, che pure sono molto importanti, ma che devono rendersi conto del fatto - - ma penso lo sappiano bene - che esiste un'attitudine, un atteggiamento molto netto da parte dell'elettorato. Tutto quel che riguarda la vicenda afghana (è chiaro che il decreto riguarda anche le altre missioni, ma noi ci concentriamo sull'Afghanistan, perché è di questo che si tratta) è inaccettabile. È inaccettabile la conferenza internazionale nel modo in cui è stata proposta, con i talebani seduti al tavolo, perché i talebani non sono gli abitanti dell'Afghanistan, non sono un'etnia, non vengono dalla città di Taleba. I talebani sono persone che hanno scelto un atteggiamento armato, un comportamento aggressivo, per i nostri *standard* terroristico, e sono i nemici di questa operazione di polizia internazionale. Pertanto, fare una conferenza internazionale sulla sicurezza dell'Afghanistan invitando i talebani sarebbe come fare una grande conferenza

In genere la nostra parte politica, il centro-destra, la *ex* Casa delle Libertà o l'attuale Casa delle Libertà - perché nell'elettorato questa sigla permane malgrado le divisioni che separano oggi i partiti al suo interno

un mito, un *cliché*, una cosa politicamente corretta, vale a dire una bugia, un'ipocrisia. Ho apprezzato molto la brutalità, più che la franchezza,

da parte della Casa Bianca, per il modo in cui l'Italia ha condotto la questione della liberazione di Daniele Mastrogiacomo. Anche in

che si trovano in giacca e maglietta, con una pistola o con fucili mitragliatori al loro fianco, senza le regole di ingaggio necessarie, senza possibilità di difendersi, senza possibilità di contrattaccare con il rischio di essere incriminati se i loro atti dovessero essere considerati da qualche sostituto procuratore della Repubblica in Italia contrari al pensiero degli stessi sostituti procuratori (perché le leggi sono molto elastiche) e quindi non sono per niente contenti. La storia per cui dobbiamo votare a favore di questo decreto-legge perché così soccorriamo i nostri soldati in Afghanistan è una balla. I nostri soldati portano un'uniforme e per questo sono obiettivi. Il ministro degli affari esteri D'Alema ha avuto l'onestà di riconoscere

visto che il nostro Governo ha delegato ad Emergency e a Gino Strada la trattativa per la liberazione (almeno è quello che è apparso) del collega Daniele Mastrogiacomo (al quale va tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà), che siamo di fronte ad una nuova visione dello Stato e degli statisti. Lo statista Gino Strada, cito il «Corriere della Sera» di martedì scorso, ha così commentato l'incarico ricevuto: «Ma che cazzo gli è venuto in mente a D'Alema di parlare di "canali umanitari". (...) Con che faccia vado a trattare laggiù? Con quella d'uno che sono sette anni che si fa un mazzo così per aiutare gli afghani e adesso si trova qui a rappresentare proprio il Governo d'un Paese che loro odiano? Io l'ho detto subito: fuori dai coglioni il SISMI, i ROS e tutti quei signori! Se hanno un capo, che li richiami subito. O noi, o loro». Questa è la nuova politica estera, questa è la dimensione civile e statale che abbiamo in quel Paese. E ho appena citato l'applauso internazionale che andiamo riscuotendo. Per questo motivo spero che anche la parte politica di cui cui sono un rappresentante cambi idea e non voti «si» a questo decreto. *(Ulivo)*. Signor Presidente, signor vice Ministro, colleghi, non può esservi dubbio che il contesto nel quale stiamo discutendo del decreto per il rifinanziamento delle nostre missioni internazionali è profondamente cambiato. Abbiamo ritirato le nostre truppe dall'Iraq, così come ci eravamo impegnati a fare; abbiamo assunto un ruolo di primo piano, e con efficacia, in Libano, evitando che la crisi apertasi nei mesi scorsi in quell'area cruciale precipitasse e si approfondisse ulteriormente; abbiamo avanzato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la proposta di una conferenza internazionale di pace sull'Afghanistan, trovando una positiva accoglienza. È assai curioso che ci si scandalizzi di fronte alla proposta, del tutto ovvia, di coinvolgere, quali parti in causa, i talebani nell'ipotizzata conferenza di pace. Con chi, se non con tutti i contendenti, occorre costruire le condizioni per porre fine, a sei anni dall'invasione statunitense, alla guerra in corso in quel Paese? Perché di guerra si tratta, come ci ricorda il rapimento di Mastrogiacomo, il ferimento del nostro paracadutista della Folgore ieri e come ha sostenuto Ban Ki Moon, segretario generale dell'ONU, sul «The Guardian» «Un numero sempre più alto di aspiranti *kamikaze* sta attraversando in questi giorni il confine tra Pakistan e Afghanistan per unirsi alla guerriglia talebana nella provincia afghana di Kandahar». Lo ha dichiarato ieri il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki Moon in una riunione del Consiglio di Sicurezza ed ha aggiunto: «Nonostante le perdite subite lo scorso anno, i talebani sembrano essersi rafforzati: negli ultimi sei mesi nel Paese ci sono stati 77 attentati suicidi, quasi tutti contro convogli militari stranieri». L'Afghanistan sta sprofondando in un nuovo Iraq, demolito nelle sue speranze, ancor più che nelle sue infrastrutture, senza riuscire ad immaginarsi una via d'uscita, dopo trent'anni di guerra senza fine e senza tregua. Lo ha sostenuto perfino il comandante britannico di ISAF. Ecco la discontinuità rivendicata sulla politica estera. È assai inquietante guardare, come hanno fatto alcuni nei loro interventi in questo dibattito, alle alle cose del mondo attraverso il proprio ombelico. La discontinuità è alla base di una ripresa di iniziative e credibilità internazionale e rende l'avvio di una seria riflessione sulle nostre missioni, sulla loro natura e sulla loro efficacia, a partire da quella in Afghanistan, del 9 marzo 2007: «L'Afghanistan è il Paese più povero del mondo. Negli ultimi anni solo il Burkina Faso e il Niger lo hanno superato nella classifica dei Paesi meno sviluppati. Dopo quasi tre decenni di guerra e un decennio di siccità, milioni di afghani non hanno ancora accesso all'acqua potabile, ai servizi igienici e all'elettricità, perfino nella capitale. Milioni di loro non ricevono cibo a sufficienza e hanno accesso, nel migliore dei casi, soltanto all'assistenza sanitaria più rudimentale. Malattie come la tubercolosi e la poliomielite, da tempo scomparse in gran parte del mondo, qui sono ancora molto diffuse e colpiscono soprattutto donne e bambini. Un bambino su quattro muore prima di raggiungere i cinque anni, per lo più a causa di malattie come il colera o la diarrea, che si potrebbero curare facilmente. La metà delle donne che perdono la vita in età fertile muore di parto: l'Afghanistan ha uno dei tassi di mortalità per parto tra i più alti del mondo. La speranza di vita media si aggira sui 42 anni. Ma le statistiche raccapriccianti non finiscono qui. Circa l'85 per cento delle donne afghane è analfabeta. Il 95 per cento di esse è sistematicamente vittima di violenze Questo è l'Afghanistan di cui parliamo. Ecco quindi le ragioni dell'aumento dei fondi a disposizione degli aiuti umanitari e della cooperazione contenuti nel decreto al nostro esame e, soprattutto, della necessità di affrontare questi nodi molto diversamente da come sinora è stato

a favore di questo decreto. Quindi, non ci dobbiamo sorprendere, ma non perché salviamo questo Governo a tutti i costi i costi (potrebbe anche essere, e alcuni hanno confermato questo, perché sicuramente quello delle destre non ci piace). Credo invece che dobbiamo salvare questa coalizione e questo Governo nel merito, anche se non su tutte le questioni siamo d'accordo.

quando bombardavano; ci sono stata con Tom Benettollo. Sono stata in tutti i territori della guerra, come donna in nero e come pacifista; ero lì quando bombardavano, so cosa sono le bombe sulla testa dei bambini, delle donne e degli uomini.

Sono questi i passaggi che mi convincono. Convincono me, che sono stata, quando nessuno era contro Milosevic

Milosevic. Dov'era l'Occidente? Allora l'Occidente era silente, non parlava dei Balcani. Dopo è venuta quella guerra, che noi non abbiamo condiviso.

ecco perché una donna pacifista può dare il consenso a queste missioni. Ringrazio per aver introdotto quel programma e quel progetto, a cui credo e spero che anche le donne dell'altra coalizione daranno sostegno. Ricordiamo che vent'anni fa, nel 1987, morì Meena, la donna che fondò Rawa, un'associazione femminista; essa fu trucidata dal KGB. Proprio in nome di quelle donne, di chi ha voluto segnare e seminare su un terreno difficile e arido; hanno seminato per poter forse, un giorno, incontrare la pace. si intende che abbia rinunciato. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà. Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, oggi discutiamo in merito alla proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali. nostri militari sono impegnati in azioni umanitarie e di interposizione nei Balcani, in Afghanistan, in Medio Oriente e in Africa, dando prova di grande solidarietà ed umanità verso le popolazioni. Hanno costruito scuole, acquedotti, ospedali, pozzi, dimostrando di essere dei veri professionisti della pace in territori dove ogni giorno si rischia la vita. Mi soffermerò, in particolare, sulla missione ISAF in Afghanistan, composta da 37 Paesi che vedono mutare gli scenari come le stagioni. Vi è una grande incertezza, un'incertezza che ho e che abbiamo riscontrato a Kabul lo scorso 9 agosto, durante la missione delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento. Un soldato, un italiano, un cittadino, in primo luogo vuole essere dal suo Stato appoggiato e sostenuto ed avere la sicurezza e sapere che si farà di tutto per tutelare la sua vita. Lo stiamo facendo? Noi riteniamo che le azioni di questo Governo non sono sufficienti. Va bene la conferenza di pace, tutta ancora da organizzare; non vi è dubbio sull'aspetto civile di questa missione, dove sono stati spesi 5,3 milioni di euro nel 2006 per sostenere con infrastrutture le popolazioni afgane. Ma dobbiamo anche considerare che la Brigata Sassari qualche giorno fa ha dovuto rispondere ad un attacco, che non siamo stati in grado di perlustrare la valle Musaquala, alle porte di Kabul, su consiglio degli americani, in quanto non adeguatamente armati per difenderci da possibili attacchi e che ieri è stato ferito un italiano in attività di perlustrazione a Farah. Sappiamo che entro poche settimane gli scontri si intensificheranno in vista dell'ormai preannunciata offensiva talebana di primavera. Ieri a New York il ministro degli esteri Massimo D'Alema ha dichiarato: «Purtroppo devo dire che la guerra, la guerriglia sta arrivando anche ad Herat e non credo che le truppe italiane siano in una buona situazione. Stiamo andando ad affrontare momenti difficili». E qui mi viene da chiedere al Governo: ma volete invitare coloro che hanno già detto di andare in guerra fra poco? Aspetterei gli eventi e poi rifletterei sull'opportunità di questa apertura nei confronti dei talebani. Il basso profilo mantenuto finora dai reparti italiani, imposto dagli equilibri politici della vostra maggioranza, non sono sufficienti a garantire la sicurezza dei nostri soldati. Mi è utile ricordare che dal 1979 al 1989 l'Armata Rossa ha perso 15.000 uomini e l'Afghanistan si è trasformato per la Russia in quello che è stato il Vietnam per gli Stati Uniti: un lungo stillicidio. È vero che i tempi sono cambiati ma la storia insegna sempre qualcosa. Non è pensabile che i nostri soldati siano dotati solo di armi di difesa passiva, ovvero una protezione fisica, segnalazione di avvisi, sorveglianza, controllo e attivazione dell'allarme. Sapete bene quanto è costato salvare la vita del giornalista Mastrogiacomo, e siamo tutti contenti di riaverlo tra noi, e allora perché non garantire massima sicurezza ai nostri soldati, che sono un esempio di volontà e di quella cultura millenaria che tutti, maggioranza e opposizione, dovrebbero con vanto esporre al mondo? L'ordine del giorno presentato dal Presidente del mio Gruppo, il senatore Schifani, e dai componenti della Commissione difesa chiede di dotare, in tempi brevi, i nostri militari di armi di difesa attiva, che non vuoi dire, come molti pensano, armi di attacco,

degli Jammer, di dotare i Puma delle torrette Hitrol. Questo perché, colleghi, la politica è importante, ma la vita dei nostri ragazzi lo è di più e non vogliamo che a causa di insicurezze interne alla maggioranza qualcuno debba pagare in termini di vita, perché ne saremmo tutti responsabili. Per questo vi chiediamo di approvare l'ordine del giorno, che consentirebbe di far vedere ai nostri soldati che ci siamo e che pensiamo e ci preoccupiamo per loro, perché questo è il primo dovere di noi tutti.

la vicenda del rapimento di Daniele Mastrogiacomo e il racconto che di quella vicenda la vittima sta facendo in questi giorni su «la Repubblica», ci dicono più di ogni altra cosa che cosa è oggi l'Afghanistan e qual è la differenza tra l'Afghanistan di Karzai e l'Afghanistan di Dudallah, tra l'Afghanistan che vuole rinascere ad una vita più pacifica e meno misera di quanto essa non sia stata per l'intero popolo nel corso della guerra dei trent'anni, che ha insanguinato e ancora insanguina il Paese, e l'Afghanistan che vuole tornare alla legge del kalashnikov e del Corano. Dai talebani Mastrogiacomo è stato incatenato, frustato, picchiato, umiliato; dai talebani ha visto sgozzare e decapitare l'autista afghano che l'accompagnava. Dal Governo Karzai Mastrogiacomo è stato invece liberato, grazie a una scelta di compromesso che è tipica delle democrazie, capaci di porre al centro dell'azione dello Stato il valore supremo della vita e della dignità dell'uomo, e non un'ideologia o un credo. È proprio delle democrazie essere capaci anche di subire la sconfitta temporanea del cedimento al ricatto, che c'è stato, pur di mantenere aperta la speranza della vittoria finale della ragione e del diritto. Karzai ha pagato un duro prezzo per aiutare un cittadino di un Paese che lo ha aiutato, e così facendo si è negato proprio a quella logica tribale che anima la violenza dei suoi nemici. Se c'è una cosa che il rapimento del giornalista italiano ci dice, dunque, è che Karzai e Dudallah pari non sono. E ci ricorda che i soldati italiani, europei, americani, australiani sono stati mandati in Afghanistan da un voto unanime del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ad interporsi tra due combattenti con uguali ragioni e uguali torti, ma ad aiutare il Governo legittimo a sconfiggere il terrorismo e l'insorgenza dei talebani; per restaurare così ordine e sicurezza nel Paese. Se è dunque opportuno e utile trattare con chiunque

quella afghana è sicuramente la più a rischio, sia per l'incolumità dei nostri soldati sia per l'esito finale della nostra azione. In Afghanistan la comunità internazionale, le democrazie del mondo, la stessa organizzazione delle Nazioni Unite sono impegnate in una sfida vitale per la pace e la stabilità dell'intero globo. La verità è che in Afghanistan noi non possiamo perdere, ma non riusciamo a vincere. È dunque del tutto legittimo e utile cercare vie nuove per vincere, a patto che sia chiaro che non possiamo perdere. Non riusciamo a vincere perché, come è chiaro ormai a tutti i *partner* della coalizione internazionale, la vittoria può essere solo politica. Non foss'altro per l'esigutà delle Forze armate impegnate in quel Paese, imparagonabile con l'impegno che è stato profuso in luoghi dove si è vinto, come i Balcani, e persino in luoghi dove non si è vinto, come l'Iraq. Ma altrettanto limitato e scarso è stato l'impegno economico per la ricostruzione di un Paese nel quale dove finiscono le strade cominciano i talebani: la miseria di 57 dollari *pro capite*. Limitato e scarso è stato il coinvolgimento degli altri Paesi della regione allo sforzo di stabilizzazione, e mi riferisco in particolare al Pakistan. Limitati e scarsi sono stati i risultati di quel lavoro di pacificazione nazionale nel quale pure il Governo Karzai è impegnato, ma senza il cui successo non è possibile dividere gli afghani dai talebani, i contadini dai trafficanti d'oppio, i *pastun* dagli studenti islamici. L'Italia, oggi membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha l'opportunità unica di far pesare adesso nelle decisioni politiche della comunità internazionale l'impegno militare che profonde in tante parti del mondo. Il nostro Governo fa dunque bene a confermare i suoi impegni internazionali e a proporsi nello stesso tempo come il motore di soluzioni nuove e creative. Su questa linea, conferma degli impegni e iniziativa politica e diplomatica per la pace, mi auguro che il Senato possa confermare quell'ampia unità nelle scelte di politica estera senza la quale un Paese non è credibile, soprattutto quando utilizza la sua forza militare fuori dai confini patrii. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia necessario stimolare la ragione in questo particolare momento, a fronte di decisioni che rischiano di essere condizionate da logiche di appartenenza partitica o da ideologie. Non intervengo dunque come senatore della maggioranza che sostiene il Governo, ma come senatore della Repubblica, come un cittadino che si considera privilegiato per avere la possibilità di esprimersi in quest'Aula. Intervengo al di fuori delle logiche partitiche cercando di portare un contributo neutro, che vuole essere di stimolo alle coscienze, nell'obbiettivo di concorrere ad una decisione ponderata che sia presa nell'interesse dell'Italia, della sicurezza e dell'operatività dei nostri militari impegnati nelle aree di crisi, delle garanzia dei diritti umani, dei diritti dei popoli, dello sviluppo della democrazia. La partecipazione dell'Italia alle missioni di pace, sulla cui riconduzione per tutto il 2007 dobbiamo esprimerci, è certamente una questione di grande importanza: non lo è perché l'esito del voto potrebbe influenzare le sorti del Governo o comunque alimentare le speculazioni sulla sua stabilità, lo è perché gli interessi in gioco, quelli veri, sono enormi. Mi riferisco, innanzitutto, alla situazione dei nostri militari impegnati nelle aree di crisi, alla possibilità di intervenire a garanzia del rispetto dei diritti umani, alla capacità di contrastare il terrorismo internazionale attraverso la diffusione della democrazia e del generale miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che vivono in quei Paesi, Paesi, alla credibilità dell'Italia sulla scena internazionale e nel quadro dell'ONU, della NATO e dell'Unione Europea. L'Italia consacra un impegno significativo nell'ambito delle missioni internazionali in atto. Non lo fa per imposizione o perché sia asservita a logiche imperialistiche o guerrafondaie, ma per una scelta assunta con coerenza e nel rispetto degli obiettivi condivisi e decisi in seno all'ONU, alla NATO e all'Unione Europea. L'obiettivo è quello di garantire la democrazia, lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto dei popoli, il rispetto delle loro culture, del loro modo di essere, delle loro peculiarità. L'intento è quello di creare e favorire le condizioni perché la pace si realizzi, affinché la stabilizzazione delle aree di tensione, l'eradicazione del terrorismo e dei germi di cui si alimenta siano la garanzia anche per il nostro stesso sistema democratico e di libertà in Italia e in Europa. Si impegnano notevoli risorse per gli aiuti umanitari e si inviano militari, donne e uomini che per il supremo obiettivo della pace e del rispetto dei diritti umani sacrificano i loro affetti e mettono a repentaglio quotidianamente vita. Il deterrente della forza non è forse quello che meglio convoglia un messaggio di pace e democrazia. Certamente, l'invio massiccio di aiuti e la realizzazione di opere umanitarie nelle aree in crisi sarebbe forse più consono, ma non è purtroppo sufficiente, perché non vi sarebbero sufficienti garanzie, in assenza di pace e democrazia, che tali aiuti intervengano in favore della popolazione civile siano invece di sostegno a quelle frange che vogliono cancellare la libertà, che alimentano il terrore e il terrorismo. Una soluzione politica e diplomatica della crisi sarebbe decisamente più auspicabile, di nuovo, ne devono sussistere le condizioni, deve esserci la possibilità di instaurare un dialogo costruttivo, non sempre possibile in presenza di condizioni di instabilità, di fanatismo, di violenza diffusa. Tra tutte le missioni, quella che desta più preoccupazioni è sicuramente, ad oggi, quella in Afghanistan, dove sono presenti quasi 2.000 dei nostri militari, in un Paese dove la democrazia sta muovendo deboli e incerti passi, grazie anche all'intervento deciso in sede ONU. Si teme però una recrudescenza, una nuova

lo ricordo - nel rispetto della Costituzione repubblicana e sotto l'egida delle Nazioni Unite, potrebbe non essere la soluzione più opportuna per favorire la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Per questo, la nostra scelta e il nostro voto sono importanti, perché ne va della nostra credibilità internazionale, ne va dell'ottenimento del risultato che avremmo voluto raggiungere con la nostra partecipazione alle missioni. Ma se la scelta sarà di continuare ad operare anche in Afghanistan, dovrà e deve essere una scelta chiara, senza pregiudizi, di pieno sostegno politico e morale: lo dobbiamo ai nostri militari per la loro sicurezza e come riconoscimento del loro sacrificio e del loro impegno. A questa scelta si dovrà comunque affiancare con determinazione la ricerca di una via diplomatica e politica, per la chiusura della crisi, anche attraverso l'organizzazione di una conferenza internazionale per l'Afghanistan che conduca alla pacificazione di quel Paese e ad un equilibrio diffuso in tutta la Regione.

Signor Presidente, i fatti avvenuti in queste giornate (il sequestro e poi la liberazione del giornalista Mastrogiacomo, il ferimento del militare italiano) e più in generale l'aumento delle azioni militari, ci confermano che la situazione in Afghanistan tende ad aggravarsi. In merito alla liberazione del giornalista Mastrogiacomo, esprimiamo il nostro apprezzamento per il risultato conseguito dell'azione del Governo e, in particolare, per il contributo di Gino Strada che, anche in quest'occasione, ha dimostrato quanto sia prezioso il lavoro che svolge in quel Paese. nonostante la situazione stia peggiorando di anno in anno, il Governo degli Stati Uniti non solo ritiene di continuare su questa strada, ma pensa di risolvere la situazione aumentando la presenza militare e gli attacchi alla guerriglia. È un'azione suicida quale conclusione porti questa politica lo vediamo non solo in Afghanistan ma anche in Iraq. Il fatto incredibile è che ci siano ancora forze politiche nel nostro Paese che non riconoscano il vero e proprio disastro che la politica estera statunitense ha provocato nel mondo. queste forze politiche, che ogni volta che manifestiamo contro la guerra ci accusano di antiamericanismo, si pronunciassero su alcuni fatti. è vero o no che la guerra contro l'Iraq è stata costruita su una montagna di menzogne, a partire dalle armi di distruzione di massa, che non sono mai state trovate e dal collegamento tra Saddam Hussein e Bin Laden, che non è mai stato dimostrato? dimostrato? È vero o no che a tre anni e oltre dalla fine della guerra il Paese è devastato, le varie etnie sono in guerra tra loro e ogni giorno, in attentati e azioni militari, perdono la vita decine e decine di persone innocenti? È vero o no che la guerra, che avrebbe dovuto portare la democrazia, ha prodotto il carcere di Abu Ghraib con le sue torture atroci e un Governo che, attraverso processi farsa, elimina con l'impiccagione i dirigenti del passato regime? regime? È vero o no che quando Saddam Hussein faceva comodo alla politica estera americana contro l'Iran è stato sostenuto, finanziato e armato dagli Stati Uniti? Uniti? Non raccontateci storie, allora, sulla lotta contro i dittatori, poiché questa non può avvenire secondo le proprie convenienze, a corrente alternata. o no, inoltre, che queste guerre, che dovevano servire a combattere il terrorismo, hanno provocato reazioni tali per cui il terrorismo - ma anche forme di guerriglia e di resistenza - si sono diffuse in modo esponenziale? Lo stesso discorso vale per l'Afghanistan. Nel corso del 2006 le vittime civili sono state 6.000, il triplo rispetto al 2005 e molte di più rispetto alla somma di tutti i morti causati dal conflitto a partire dal 2002.

I talebani controllano il Sud e l'Est del Paese e la loro iniziativa sta penetrando ad Ovest e nella capitale, dove sono presenti i militari italiani. La produzione dell'oppio è aumentata come non mai e copre il 90 per cento della produzione mondiale. Di fronte a questi incontestabili fatti, come si fa a non prendere atto di un vero e proprio fallimento della propria azione e a non cambiare radicalmente linea? La verità è è che le motivazioni vere di queste guerre, sia di quella irachena che di quella afghana, non c'entrano nulla né con la lotta al terrorismo, né con l'esportazione della democrazia. Il controllo di zone ricche di risorse energetiche, come l'Iraq, o di Paesi che, come l'Afghanistan, si trovano a ridosso delle nuove potenze emergenti (Cina, India e Russia) sono le motivazioni vere di queste guerre. Gli Stati Uniti hanno bisogno di tutto questo per tenere in piedi un'economia che viaggia ben al di sopra delle proprie possibilità. Il nostro Paese non ha alcun interesse a seguire questa politica. Il Governo precedente si era legato mani e piedi a tutte le scelte dell'Amministrazione Bush, ma il nostro Governo deve operare

e voterò comunque come decide il mio Gruppo - che la soluzione migliore sia quella di calendarizzare il ritiro dei militari italiani dall'Afghanistan, praticare una politica di pace e di riduzione delle spese militari, non consentire il raddoppio della base di Vicenza e lavorerò insieme al Movimento per la pace perché questi obiettivi si realizzino. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ormai questa vicenda si stia trascinando con grande fatica. Vorrei partire dalle dichiarazioni del ministro degli affari esteri D'Alema, rese ieri sera al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché di polemiche ne abbiamo fatte molte. Noi di Alleanza Nazionale, che con grande tormento ci stiamo avviando a decidere come voteremo (non è scontato il nostro voto favorevole), vorremmo cercare almeno di mettere alcuni punti fermi sulle cose che da oggi in poi dobbiamo fare. pronunciato una dichiarazione importante; ha affermato che la sicurezza in Afghanistan è la priorità per la stabilità del Governo Karzai. Apprezziamo questa dichiarazione.

nel rimettere in discussione, o perlomeno capire, se i *caveat* entro cui operano le truppe italiane sono ancora validi, non solo quelli relativi alle regole di ingaggio

alle aree che abbiamo definito oltre le quali i soldati italiani non entreranno in azione. Ci domandiamo, cioè, se nel momento in cui nella zona di Farah, quindi al confine della provincia di Herat, i soldati italiani saranno impegnati ed autorizzati a sparare (perché, evidentemente, se verranno aggrediti da talebani in fuga saranno autorizzati a compiere questo tipo di azioni), questo evento che si prospetta come ragionevole (lo ha detto lo stesso ministro D'Alema al termine delle sue dichiarazioni presso il Consiglio di Sicurezza) non debba essere oggetto di discussione. Il vice ministro Intini ieri sera ha dichiarato giustamente, anche lui, che la politica stabilisce degli obiettivi e sono poi i militari a decidere se i mezzi a disposizione delle forze italiane sono sufficienti per svolgere i ruoli. Noi ribadiamo che la politica deve riflettere e ridefinire la posizione delle truppe italiane all'interno dell'ISAF e nei rapporti con gli altri *partner* della NATO e con gli Stati Uniti ed è in funzione di questa riflessione, di questa decisione, di questa conferma, alla luce anche delle nuove situazioni di attacchi preventivi condotti dalla NATO per garantire la sicurezza in Afghanistan, che saranno date le opportune disposizioni della politica alla difesa e saranno poi i militari a stabilire di quali armi hanno bisogno, anche se - noi ne siamo convinti - oggi non sono messi in condizioni di operare al meglio. corso una polemica con il senatore Furio Colombo sul fatto che si debbano leggere sempre i giornali americani per capire cosa succede in Italia, opinione peraltro assai discutibile. Io non leggo i giornali americani, ma le agenzie che provengono dagli Stati Uniti,

Gli USA hanno definito pessima l'idea di invitare i talebani alla conferenza, hanno dichiarato che sono stati liberati cinque talebani molto pericolosi

perché ho troppa stima dell'onorevole Fassino per pensare che la sua dichiarazione sia stata un incidente di percorso. Probabilmente, il segretario dei DS si è sacrificato in questa vicenda per fare un'apertura che il Governo non poteva fare, per garantire in questo momento ai talebani che da parte del Governo italiano - o almeno delle forze politiche di maggioranza - si sarebbe prestata una particolare attenzione.

ha in animo di fare e fa per rafforzare le istituzioni in Afghanistan). Ne ha riproposta una, secondo noi fuori tempo, perché una Conferenza internazionale di questo tipo non ha senso senza il Pakistan; forse, il ministro D'Alema,

percorsi e *Road Map* - anche se portano spesso sfortuna - in politica bisogna stare attenti ai tempi: non è detto che le idee giuste, collocate in tempi sbagliati, siano politicamente corrette. Riteniamo, infatti, che la Conferenza internazionale possa avere una propria validità,

telefonato al Primo ministro dell'ANP (l'Autorità Nazionale Palestinese) garantendo ciò che non si può garantire, anche perché tutto il mondo e la comunità internazionale riconoscono che il nuovo Governo dell'ANP non ha ottemperato a una prima richiesta,

censura. Non è possibile che anche su questo fronte l'Italia si smarchi nei confronti di un Presidente dell'ANP che, prima di tutto, sta dimostrando di essere *leader* di Hamas piuttosto che uomo di Governo del futuro Stato palestinese. Un'altra osservazione riguarda i Balcani.

Abbiamo però l'occasione dei Balcani, che sono in Europa, appartengono e apparterranno all'Europa. Stiamo lavorando per farli entrare nell'Unione Europea. In quell'area l'Italia deve avere un ruolo da protagonista, perché è la più vicina a quel punto di crisi, e deve dimostrare la sua capacità

In occasione di quel dibattito, che fu molto acceso, la questione esaminata in maniera dirimente fu quella relativa al fatto che il Governo decise, a nostro avviso sbagliando, impropriamente, di porre la questione di fiducia. Noi dicemmo, con grande chiarezza, che non c'erano i motivi per la fiducia. Assumersi la responsabilità di porre la questione di fiducia su questioni di politica estera è un errore madornale.

avrebbe diviso il Parlamento e testimoniato così che il nostro Paese non aveva l'autorevolezza e la compattezza per sostenere queste missioni militari. Ebbene, in quell'occasione prevalse una volontà diversa e io sono qui a rileggere le parole con le quali la Capogruppo dell'Unione sostenne

». Allora, chiedo alla collega Finocchiaro: ha cambiato idea? È successo qualcosa di diverso? C'è stato qualche elemento che

la questione di fiducia e oggi non lo fa più? Ditelo! Ditelo con chiarezza: lo fate perché allora per voi era indispensabile dimostrare l'autosufficienza dei voti sulle questioni di politica estera e oggi non potete più farlo perché siete sicuri di non avere più l'autosufficienza. Non avete più l'autosufficienza! Non lo dico perché è un'opinione espressa così, senza un dato concreto; lo dico perché il Senato ha dimostrato che, sulle questioni di politica estera, il Governo non ha la maggioranza. Non ce l'avete! Dovete prenderne atto. E fareste bene, in maniera responsabile, non solo a prenderne atto, ma anche ad evitare di perseguire un obiettivo che è solo quello di durare e di mantenere il potere politico. Questo non è governare, questo è durare, questo è sopravvivere, questo è utilizzare *escamotage*, trucchi ed espedienti,

Pensate che non sia evidente, palese, sotto gli occhi di tutti, che non ci sono i voti, che non c'è l'autosufficienza? Suvvia, chiedo a voi uno scatto di orgoglio nel dire: «Va bene, riconosciamo che questa è la situazione; prima che sia troppo tardi, lo riconosciamo».

esiziali per il Paese. Dimostrate quindi di voler durare, di voler non governare, ma sopravvivere, di arrampicarvi sugli specchi, cercando di mettere d'accordo tutti, il diavolo e l'acqua santa. E per farlo utilizzate anche espedienti dialettici. Il segretario

Al di là del fatto che già sui tempi si potrebbe discutere, perché una conferenza di pace non si organizza dall'oggi al domani, nel frattempo però i soldati andrebbero sostenuti in questa loro presenza

All'interno della vostra stessa maggioranza, il collega Polito qualche minuto fa ha avuto modo di dire che non è neanche possibile immaginare una cosa del genere. Quindi, desidero chiedere al Governo

Smentite il vostro segretario nazionale? Smentitelo, perché questo succederà, oppure il Governo affermi che la linea politica è fare una conferenza di pace con i talebani. Ma delle due l'una. Non esiste una terza possibilità e qualsiasi strada sceglierete dimostrerà che il Governo non è in sintonia con uno dei partiti più importanti o che non ha il sostegno di questi partiti e quindi, anche da questo punto di vista, palesate le vostre difficoltà interne.

I vostri «senza se e senza ma» cosa sono se non l'intento di mantenere il potere? Sono dei «senza se e senza ma» indipendentemente da ciò che succede: restare e sopravvivere. Spiegatelo a quelli che prendete in giro quotidianamente che i vostri «senza se e senza ma»

Quale senso di responsabilità è il vostro nel dire non sono d'accordo ma voto sì pur di stare a galla e mantenere il Governo, rispettoal nostro che avremmo tutto il titolo dal punto di vista politico nel dire votiamo «no» perché voi non avete la maggioranza? Nonlo facciamo - contrariamente a quanto ci avete accusato di fare in maniera strumentale - perché mettiamo davanti l'interesse generale del Paese al nostro interesse. Infatti, se l'interesse fosse solo politico con il nostro voto negativo andreste a casa; quindi è solo il senso di responsabilità che ci impone di privilegiare l'interesse del Paese a quello specifico e personale. Voi, invece, fate il contrario. Questo è il vostro senso di responsabilità. Non si governa un Paese così, cari amici. Non si governa un Paese importante come l'Italia con questi mezzucci e con questi atteggiamenti e spero che chi - sono convinto ve ne siano tanti al vostro interno - ha ancora il senso dello Stato, dell'istituzione e della politica rifletterà, perché questa è una strada sbagliata.

dopo l'Afghanistan e dopo l'Iraq, limiti e risultati del contrasto al terrorismo emergono con qualche chiarezza. In particolare emerge un insegnamento: tutte le dimensioni dello spettro d'azione della comunità internazionale sono necessarie ed inscindibili, quella diplomatica, quella militare e quella economica. Dunque, Conferenza di pace, conferma dell'impegno militare, accentuazione dell'impegno economico e umanitario. In tal senso già nella titolazione del provvedimento in esame si evidenzia una sostanziale correzione. L'intero titolo primo è dedicato agli interventi di cooperazione, sviluppo e di carattere umanitario. E quale maggiore impegno politico della comunità internazionale ci può essere di una conferenza di pace sulla quale l'Italia sta lavorando in sede europea, alle Nazioni Unite e con gli Stati Uniti, nostro principale Paese amico e alleato, ritrovando in ciascuno di questi attenzione, sostegno e condivisione? Collega Antonione, non c'è niente da smentire. Spetta al Governo di Kabul, non certo alla polemica politica italiana - come ha ricordato il ministro D'Alema - decidere chi debba partecipare alla Conferenza sul futuro dell'Afghanistan, ben sapendo che il presidente Karzai ha proposto un programma di riconciliazione rivolto a chi accetta di rinunciare alla guerra deponendo le armi per partecipare al processo democratico. In questo contesto credo vada evitato il rischio del pendolo, vale a dire che si vada da un estremo all'altro, dall'accentuazione di un impegno in sola chiave militare (come sembra di sentire da certi interventi in questo nostro dibattito) al suo opposto, ad un disimpegno, che già il legittimo Governo afghano ci ha chiesto di scongiurare. La necessità di una dimensione militare non va banalizzata, per il pericolo che uno squilibrio militare sul campo a favore delle milizie antigovernative, contro un Governo insediatosi dopo libere elezioni democratiche, possa rendere vana la dimensione diplomatica e quella di ricostruzione economica e sociale. A tale proposito, mi chiedo che utilità abbia rappresentare un quadro non veritiero dell'impegno dei nostri militari per la sicurezza a Kabul ed Herat, definito e concordato non unilateralmente, ma in ambito NATO ed in epoca precedente a quella attuale, vale a dire nella scorsa legislatura, da altra maggioranza, da altro Governo. Dunque, questa specie di corsa, un po' schizofrenica, ad una sorta di *diminutio* del lavoro del nostro contingente non ha alcun fondamento reale. Tuttavia, rischia di svilire oltre che il sacrificio e la professionalità delle nostre forze armate, il contributo che l'Italia dà ad una missione impegnativa, difficile e rischiosa, per la quale siamo ad un tempo grati alle Forze armate ed orgogliosi degli uomini e delle donne che le compongono, non meno di quanto lo siamo per l'impegno dei nostri e delle

Fin dalla risoluzione delle Nazioni Unite 1386 del dicembre 2001, ISAF ha il compito di garantire la sicurezza di autorità afghane e di assisterle nel perseguimento di una cornice di sicurezza indispensabile alla pacificazione e ricostruzione dell'Afghanistan. In una prima fase questo impegno è stato limitato a Kabul. Successivamente, in cooperazione con le ricostruite forze di sicurezza afghane, questo impegno si è esteso, attraverso i PRT, in varie province, ad una rilevante parte del territorio. Ricordo che quando si decise questa estensione di impegno, coincidente con l'assunzione del comando ISAF da parte dell'Alleanza atlantica, un notevole scetticismo accompagnò anche in quest'Aula quella scelta. Si disse che oltre Kabul non era possibile andare. I fatti dimostrano il contrario, come ha potuto constatare la delegazione di Senato e Camera ad Herat. L'attività di ricostruzione e sviluppo dei servizi, particolarmente nel settore scolastico e socio‑sanitario, delle infrastrutture e delle istituzioni, ha realizzato significativi progressi. Ha fatto intravedere a quelle popolazioni altre opportunità possibili, realizzabili, in un quadro di sicurezza. Quella sicurezza indubitabilmente accresciuta rispetto alla condizione pre-ISAF ad Herat e Kabul. Certo, anche da questo punto di vista non vanno sottovalutati i pericoli di una possibile accentuazione dei rischi. E a tale proposito ritengo bene facciano il Governo e la maggioranza a non escludere aprioristicamente l'eventualità di adeguare le originarie regole di ingaggio ed il relativo e conseguente assetto sul campo ove mutasse la cornice di sicurezza attualmente in essere. Per ora non ci sarà un cambiamento dei criteri di impiego, delle regole di ingaggio, della dislocazione territoriale. Ci sarà, però, un aumento della protezione passiva del nostro contingente, dotandolo dei nuovi veicoli a maggiore resistenza ad attacchi esplosivi, così come una maggiore capacità di sorveglianza del territorio grazie ai velivoli senza pilota. Signor Presidente, colleghi, le altre missioni non sono meno rilevanti e impegnative, quali quelle UNIFIL in Libano. Vorrei ricordare a qualche collega che mi ha preceduto che la risoluzione delle Nazioni Unite relativa alla missione UNIFIL non prevede affatto, tra i compiti del nostro contingente, quello di disarmare Hezbollah. Quando si sentono in quest'Aula simili affermazioni, c'è da chiedersi se siano state adeguatamente lette le disposizioni che hanno portato il nostro Paese a impegnarsi in quella missione.

liberando da ragioni riconducibili alla polemica politica interna le determinazioni circa l'impegno del nostro Paese in ambito internazionale. Tale impegno è svolto nel quadro di una solida alleanza con gli Stati Uniti, oltre che in coerenza con i tre pilastri fondamentali della nostra politica estera: le Nazioni Unite, l'Europa e l'Alleanza Atlantica.

a un adeguamento degli *standard* di sicurezza di fronte a un eventuale modificarsi della situazione sul campo. Del resto, abbiamo piena fiducia nei comandi militari, nella loro professionalità - ormai largamente collaudata da anni di esperienza di missioni in aree a rischio - e la politica è pronta a dare risposte adeguate alle eventuali richieste dei comandi militari. Diverso è invece il discorso sull'ipotesi che si possa procedere a una *escalation* dell'impegno militare del nostro Paese e dei nostri alleati che miri a una sorta di autosufficienza della dimensione militare della missione. missione. È evidente che è un punto che va approfondito. Naturalmente, ci distinguono in quest'Aula diversi approcci di tipo culturale e politico rispetto al tema delicatissimo dell'uso della forza,

è piuttosto difficile immaginare di controllare un territorio vasto e impervio come quello dell'Afghanistan ed è impossibile pensare di controllare in maniera stabile persino soltanto la linea di confine tra Afghanistan e Pakistan. Per questo occorre una soluzione politica ed è per questo che il nostro Governo è impegnato con la proposta della conferenza internazionale che deve coinvolgere gli altri attori della Regione e ricercare, insieme ai nostri alleati ma, innanzitutto, assieme al Governo Karzai, una soluzione politica di stabilizzazione dell'Afghanistan. Su questo credo che il Parlamento possa trovarsi unito. Concludo con una battuta sulla questione della fiducia e dell'autosufficienza. Sono, colleghi, due facce della stessa medaglia. Non ho nessuna difficoltà

un errore porre la questione di fiducia su un tema così delicato come la presenza dei nostri militari all'estero. L'ho detto in quella circostanza e non ho difficoltà a ripeterlo. Tuttavia, l'apposizione della questione di fiducia non è che l'altra faccia della campagna sull'autosufficienza. Ora, credo che non esista paese del mondo occidentale nel quale la maggioranza pone la fiducia sulla presenza dei militari all'estero, ma non esiste neanche Parlamento al mondo nel quale l'opposizione sfida la maggioranza circa la propria autosufficienza su una materia come questa*.* Altrimenti il Governo Blair, in occasione dell'intervento in Iraq, avrebbe dovuto dare le dimissioni e tornare al voto.

gli schieramenti si arrivasse a considerare positiva la convergenza parlamentare su un tema così vitale com'è la nostra proiezione sulla politica estera, credo che la nostra democrazia farebbe un passo in avanti. *relatore*. Signor Presidente, se dalla discussione in cui sono intervenuti più di 30 senatori si scomputano i toni e gli argomenti dialettici, la sintesi che se ne può trarre segna una convergenza sostanziale più ampia di quella che presumibilmente si leggerà domani nelle cronache dei giornali, o magari già questa sera negli intrattenimenti televisivi. Vi è convergenza sostanziale circa il fatto che la partecipazione italiana alle missioni internazionali debba continuare per gli scopi cui è finalizzata e che i militari in essa impegnati siano dotati di regole, mezzi ed armi proporzionati al compito, comparabili con gli altri Stati che che concorrono alle iniziative multilaterali, adeguati alla protezione delle popolazioni nei territori che sono segnati sulle mappe dal tricolore nazionale. In particolare, per l'Afghanistan, che al momento è il punto più caldo sulla mappa dei rischi, l'attuazione da dedicare agli armamenti del contingente italiano è un imperativo cui certamente il Governo non vorrà sottrarsi e di cui il Parlamento dovrà essere costantemente e puntualmente informato. Il termine ormai imminente della conversione del decreto rende di fatto impraticabili gli emendamenti, che comporterebbero il rinvio alla Camera. Ma negli ordini del giorno, presentati da tutti i Gruppi, si trovano elementi di riflessione che credo debbano essere considerati con attitudine aperta e positiva.

Mi pare ci sia stato un approfondimento importante e che nonostante le molte polemiche, come ha osservato il senatore Zanone, ci sia una sostanziale unità sui princìpi base della nostra politica estera. Si è parlato quasi soltanto di Afghanistan, anche se le missioni sono una ventina, anche se quella afghana non è la più numerosa e neanche quella in cui l'Italia ha le maggiori responsabilità: il Libano è per noi l'impegno più importante. Tuttavia tutto ciò è naturale, perché oggi l'Afghanistan è al centro, in modo drammatico, delle preoccupazioni dell'opinione pubblica. Voglio fare una riflessione: storicamente la crisi dell'Afghanistan somiglia a quella dei Balcani. Tutte e due vanno avanti da un secolo e mezzo, le nostre generazioni erano disinformate su entrambe,

nei Balcani come in Afghanistan, si sono scaricate le tensioni fra tre grandi attori globali: la Russia, l'Islam e l'Occidente. Questo era quello che in Afghanistan veniva chiamato nell'Ottocento dagli inglesi il *big game*, la grande partita, quello che i generali zaristi chiamavano il torneo degli spettri tutti chiamavano il buco nero. Il buco nero che assorbiva e faceva sparire gli eserciti: il buco nero ha divorato gli inglesi e ha divorato gli eserciti gli eserciti russi. Noi vorremmo salvarci, anche perché non vogliamo affermare un impero, non rappresentiamo una nazione, ma le Nazioni Unite. Vogliamo soltanto evitare che il buco nero getti la sua ombra su New York o su Roma, proiettando verso di noi gli spettri del nostro tempo, cioè i terroristi islamici. Faccio questo parallelismo con la crisi dei Balcani non per caso. Chi ha stabilizzato i Balcani? Innanzitutto i Paesi vicini: ci stupiremmo se nei Balcani agissero i Paesi asiatici e l'Europa fosse completamente assente. Bene: i Paesi confinanti con l'Afghanistan devono dare il loro contributo, anche perché hanno tante chiavi per agire sul terreno afghano. Questa è, nella sostanza, la logica di una Conferenza internazionale. È una nostra proposta, non si realizzerà domani, ma raccoglie crescenti consensi e questo dovrebbe essere considerato positivo dalla maggioranza e dall'opposizione. Hanno un peso i Paesi confinanti in Afghanistan? Certamente sì. Hanno interessi forti e spesso contrastanti? Sì. Si mettano dunque le carte in tavola, si affrontino i nodi politici, perché l'azione militare è necessaria ma non sufficiente. Il Pakistan è il santuario dei guerriglieri talebani ed è il tutore dell'etnia afghana pastun comune a parte del Pakistan stesso. Nella Kabul dei talebani c'erano tre ambasciate: quella saudita, quella degli Emirati e quella pakistana e l'ambasciatore del Pakistan era chiamato il viceré. L'Afghanistan destabilizza con il suo fondamentalismo il Pakistan. Musharraf è probabilmente leale, ma trova una formidabile opposizione islamica filotalebana nel suo stesso Paese. L'India ha sempre appoggiato, contro i pastun, l'alleanza del Nord guidata dai tagiki e teme che l'Afghanistan destabilizzi con i suoi fondamentalisti islamici il Kashmir musulmano. Pakistan e India, non dimentichiamolo, sono due potenze nucleari che si contrappongono in Afghanistan. La Russia vede le Repubbliche ex sovietiche e se stessa minacciate dall'infezione fondamentalista islamica esplosa in Afghanistan. Anche per questo ha avuto decine di migliaia di morti, in una lunga guerra, che forse non era dettata soltanto da mire imperialiste. La Cina ha lo stesso problema: un'opposizione fondamentalista islamica e separatista legata all'Afghanistan nella sua provincia dello Xinjiang. L'Iran è il nemico storico dei talebani sunniti, difende le sue minoranze sciite in Afghanistan ed è invaso dalla droga proveniente dall'Afghanistan, che provoca decine di morti. Pakistan, India, Cina, Iran e Repubbliche ex sovietiche devono dunque mettere con noi le carte in tavola. Possono dare un aiuto decisivo, naturalmente se il Governo Karzai è d'accordo. Se una Conferenza internazionale aprirà la strada, se le condizioni lo consentiranno, il Governo Karzai vorrà in futuro sedere ad un tavolo anche con i talebani? Io credo di sì ed è quasi ovvio. Il Governo Karzai conosce i talebani meglio di noi, sa che sotto quella etichetta ci sono almeno quattro diverse realtà: i terroristi, i narcotrafficanti, i capi tribali e i capi religiosi. Vuole dividere, non unire i suoi e i nostri I terroristi vanno distrutti, con i capi tribali si è sempre trattato. Molti che erano capi talebani oggi siedono in Parlamento. Io stesso ho trattato nel 2001 con il ministro degli affari esteri talebano Mutawakil, che oggi sta nel sistema politico legale afghano. La pace si fa non uccidendo tutti i combattenti nemici, ma facendo loro deporre le armi. Da sempre questo è l'abc. Il Governo Karzai d'altronde ha proposto l'amnistia per tutti i crimini orrendi degli ultimi trent'anni, purché appunto si depongano le armi. Questa è la strada politica che deve accompagnare quella militare. Sull'impegno militare parlerà il sottosegretario Forcieri

in Italia e solo in Italia si deve chiedere all'Italia e soltanto all'Italia di fare qualcosa di più e di diverso di quello che si chiede ai nostri alleati europei della NATO? Qualcuno dice che occorrono più soldati, ma l'Italia ha il quarto contingente, dal punto di vista numerico, in Afghanistan e largamente il primo in Libano. E perché si deve chiedere all'Italia un impegno immensamente superiore al suo peso in campo internazionale? L'impegno militare non basta mai, però è spesso un aiuto. In Afghanistan, ad esempio, ha aiutato, in Iraq no. Questo va detto. L'Afghanistan non è l'Iraq, non soltanto perché in Afghanistan c'è il multilateralismo e in Iraq c'è stato un esempio di unilateralismo, ma per ragioni più concrete. L'Afghanistan non è soltanto una storia di fallimenti ed i fatti pesano: in Iraq 2 milioni di cittadini se ne sono andati in esilio all'estero, in Afghanistan 4 milioni e mezzo sono tornati; in Iraq il 50 per cento dei bambini non va più a scuola, in Afghanistan 7 milioni di bambini sono tornati a scuola.

Voglio fare in proposito una semplice considerazione: Israele per vent'anni ha occupato il Sud del Libano e, nel frattempo, Hezbollah si è armata come ben sappiamo.

delle armi. Anche in Palestina e in Libano la politica sarà decisiva: la guerra in Libano è finita grazie all'impegno dell'UNIFIL, ma questo è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Il processo di pace si deve allargare alla Palestina e presto, altrimenti la crisi palestinese incendierà di nuovo anche il Libano. Il Governo di unità nazionale in Palestina è un passo avanti: la comunità internazionale, da un lato, insisterà perché esso adempia pienamente alle richieste del quartetto che comportano anche il chiaro riconoscimento d'Israele; dall'altra parte, la comunità internazionale cercherà di non sciupare l'opportunità che questo Governo può offrire per l'apertura di un negoziato. In conclusione,

definito un multilateralismo efficace, sotto l'egida delle organizzazioni internazionali (le Nazioni Unite, l'Unione Europea e la NATO) e nel pieno rispetto dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Le nostre missioni ora, chiuso quello che è stato il *vulnus* pesante dell'Iraq, corrispondono tutte a queste caratteristiche: legittimazione internazionale, ampia partecipazione dei Paesi soprattutto europei, quindi ampia multilateralità, finalità e motivazioni a scopi pacifici. Si è parlato in particolare dell'Afghanistan.

degli aspetti che caratterizzano questa missione. È una questione sicuramente importante che riguarda la sicurezza, ma l'impegno della comunità internazionale in quell'area, in quel Paese è molto più ampio, riferendosi a tutti quei processi di *Nation* *building* che comportano interventi di carattere civile, economico e politico. Non a caso tre sono gli obiettivi della comunità internazionale: la sicurezza, la formazione di uno Stato di diritto nel rispetto dei diritti umani e lo sviluppo economico di quel Paese. Sono e siamo tutti ben consapevoli che non è attraverso la sola dimensione militare che si può arrivare ad una soluzione per questi problemi e per questo Paese. Credo però sia giusto, anche aiutato dalle ampie considerazioni di carattere politico generale svolte dal collega Intini, che io mi soffermi soprattutto sulle questioni di carattere militare, sollevate militare, sollevate da molti oratori, a partire da quelle citate dal presidente Cossiga, che ha addirittura ipotizzato uno sganciamento dalla NATO e dal comando ISAF e la trasformazione di una missione militare in una missione umanitaria, citando i nostri interventi nel settore civile. A me dispiace che si sia affrontato questo tema con, a mio giudizio, un eccesso di ironia e, quindi, con un eccessivo carico polemico. l'aspetto della collaborazione civile e militare nelle missioni internazionali sta ormai diventando, anzi è diventato parte integrante della missione. Credo che noi dovremmo rilevare tutti con orgoglio come un particolare modo di operare dei nostri militari, soprattutto nel rapporto con le popolazioni civili, sia diventato prima oggetto di materia di insegnamento anche nelle scuole militari di di altri Paesi e di Paesi anche grandi - mi riferisco alla scuola militare dei *marines* negli Stati Uniti d'America - e poi un concreto comportamento pratico di tutte le forze militari occidentali che operano nelle missioni internazionali, a partire da quelle dei Paesi NATO. Oggi la cosiddetta SIMIC, la cooperazione civile e militare, rientra in tutte le pianificazioni di carattere militare delle nostre Forze armate, così come di quelle dei Paesi NATO ed europei. È assolutamente importante, cioè, per il buon successo dell'operazione che l'aspetto della sicurezza non sia disgiunto, ma anzi sia strettamente connesso al consenso delle popolazioni

che però vanno incontro a problemi ed esigenze reali di quelle popolazioni, creano un sistema di fiducia e, alla fine, secondo me, rappresentano alcuni dei motivi che possono garantire il successo delle nostre delle nostre operazioni. Non è un caso se nelle settimane scorse proprio uno dei più prestigiosi giornali americani, «The Washington Post», ha pubblicato un articolo di un corrispondente da quelle zone intitolato «Nella valle afghana, una guerra pacifica» cui si affermava che fonti ufficiali dicono che l'opera delle truppe italiane, così come quella degli altri, che forniscono sicurezza, addestramento, assistenza e sviluppo alle aree povere e potenzialmente ostili dell'Afghanistan, può essere più efficace delle sortite militari, che talvolta irrompono nelle case, fanno vittime e, quindi, possono alienare le comunità locali. Di questo si tratta, di una precisa politica che fa parte ormai della nostra pianificazione militare (per «nostra» intendo di tutti i Paesi che fanno parte della NATO). Si è discusso delle questioni che riguardano le regole d'ingaggio, i *caveat* e le attrezzature e gli equipaggiamenti dei nostri militari. Circa le regole d'ingaggio,

È chiaro che le regole d'ingaggio di tale missione sono state definite in ambito NATO, naturalmente con il consenso ed il concorso di tutti i Paesi (perché, come sapete, nel regime della NATO vige il principio dell'unanimità). Queste regole d'ingaggio corrispondono alle necessità operative che i militari devono osservare per far sì che i loro comportamenti siano coerenti tra di loro e che corrispondano all'obiettivo che si vuole raggiungere. L'autorità politica, cioè, fissa l'indirizzo; le regole d'ingaggio, poi, devono essere tali da consentire all'autorità militare di tradurre in codificazione operativa concreta e fattibile tali linee d'indirizzo.

intenzioni ostili nei nostri riguardi; nonostante ciò, è precisa volontà mia e della Difesa rendere nota al Parlamento la sostanza delle regole e i criteri dell'impiego dei nostri militari, per eliminare sia ogni perplessità reale sia ogni elemento strumentale che sul punto è stato e può essere ancora sollevato. Le regole consentono sicuramente l'elaborazione di comportamenti sicuri e chiari per quanto riguarda l'autodifesa, lasciando al comandante la possibilità di utilizzare la forza in modo adeguato alle circostanze. Quindi, se si viene attaccati o se viene riconosciuta una situazione di imminente attacco, i nostri militari dovranno e potranno difendersi in modo adeguato. Per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni, le regole consentono l'uso della forza per far rispettare gli scopi della missione: è questa, chiaramente, la parte più critica e delicata, perché impone un comportamento attivo, soggetto anche a possibili resistenze. Voglio ricordare che la missione ISAF si inquadra nell'articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite ed è una missione di *peace enforcing*, per cui prevede anche l'uso della forza: l'uso della forza: questo, infatti, sarà pienamente consentito contro chiunque tenti di impedire ai militari di rispettare i propri compiti e di limitarne la libertà di movimento; è consentito di intervenire attivamente anche nel caso venga messa in pericolo l'incolumità della popolazione civile. Pertanto, i nostri militari potranno agire con i mezzi a disposizione per impedire qualsiasi attività ostile venga effettuata nell'area di propria competenza. Vi è, quindi, piena coerenza tra gli obiettivi e gli strumenti, perché vengano messe a disposizione tutte le adeguate autorizzazioni all'uso della forza per realizzare gli scopi della missione. Data per certa l'adeguatezza delle regole d'ingaggio, è però importante precisare i criteri con cui esse saranno adottate: le regole di ingaggio, infatti, sono solo uno strumento di base; la situazione sul campo è e sarà sempre e comunque delicatissima, richiede una grande dose di freddezza e buonsenso nella loro applicazione: questo fa parte dell'addestramento e della dimostrata esperienza - che ho già richiamato - dei nostri militari. Anche da questo punto di vista, il comportamento dei nostri militari non deriva da una sorta di «italiani, brava gente», come si vuol far credere, ma da una precisa scelta che riguarda la formazione e l'addestramento, che punta ad individuare

quando possono mettere in discussione questo (il sacrificio della vita propria o altrui), costituiscono un'*extrema* *ratio* che non è mai data per scontata. Questa è una filosofia che, nel salvaguardare l'incolumità dei soldati sul campo, induce i comandanti ad un preciso autocontrollo per evitare errori ed incidenti. L'esperienza da noi maturata in queste missioni ha dimostrato

senatori disquisire sullo spessore delle nostre corazze e sull'adeguatezza dei nostri mezzi. Diffido di una politica che debba anche stabilire quale tipo di pistola, di fucile o di giubbetto antiproiettile debba avere un militare:

strumentale e polemica per voler per forza dire che le cose sono cambiate in peggio per quanto riguarda le nostre regole e i nostri equipaggiamenti: non è così, e quindi mi auguro che,

tutti siamo impegnati a dare il nostro contributo.

Tutti i provvedimenti sono importanti, però credo che più importante di tutto debba essere la vita di un decreto e la sua conversione in legge quando siamo all'ultima settimana